L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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

relazione orale e ha avuto inizio la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice La Mura. Ne ha facoltà.

L'istituzione che rappresenta i cittadini non serve più, perché, al di là dei proclami, questo Governo non sta facendo gli interessi dei cittadini; ne abbiamo consapevolezza e ci sono i fatti che parlano. Nelle settimane scorse e fino alla notte tra il 20 e il 21 dicembre, la maggioranza del Governo Draghi,

la maggioranza a porte chiuse si è appropriata per giorni della legge di bilancio, fino a quando non ha raggiunto gli accordi su tutto il pacchetto di proposte prima di votarle in un'unica seduta fiume, di notte. Ci avevano chiesto di segnalare solo due emendamenti tra tutti quelli che avevamo depositato. Anche questa prassi è consolidata, ma nella notte tra il 20 e il 21 dicembre hanno votato solo quattro fascicoli di emendamenti della maggioranza, riformulati anche sei o otto volte per ottenerne l'approvazione, facendo letteralmente morire tutti gli altri presentati, come se non fossero mai esistiti. Ieri finalmente ci hanno lasciato entrare in Commissione, solo alla fine della seduta ufficiale - pura parvenza - e hanno concesso a chi lo chiedeva di svolgere il funerale degli emendamenti che erano stati considerati morti. Sì, sembra un racconto di fantasia, ma è la realtà. Ieri, qualche minuto prima delle ore 15, ho chiesto che i miei emendamenti venissero votati, affinché ogni singolo voto contrario consentisse a ciascun emendamento di essere registrato tra quelli che troverete sul sito del Senato, per evitare che finisse nella fossa comune dei senza nome. Sapete perché l'ho fatto? Perché ogni emendamento presentato rappresenta problematiche da gestire e risolvere dei cittadini e dell'Italia. Un esempio sono gli emendamenti relativi al bacino idrografico del fiume Sarno, una piaga sociale che dura da troppo tempo (almeno cinquant'anni), perché la politica non vuole occuparsene. Ho proposto che il bacino idrografico del fiume Sarno venisse individuato come sito di interesse nazionale, considerato il degrado ambientale in cui versa e il pericolo per la salute dei cittadini e per l'economia. Il mio secondo emendamento, sempre

eppure nessuno di voi lo ha sostenuto: ne darete conto ai cittadini. Ho presentato emendamenti per rimediare all'inaccettabile situazione in cui versano i dipendenti dell'ex Corpo forestale dello Stato, la riforma Madia ha mortificato, determinando un'irragionevole dispersione di preziose competenze, soprattutto oggi che con il PNRR e la transizione ecologica abbiamo bisogno di persone competenti. Oggi prenderemo persone che non conoscono il territorio. Inoltre, bisogna rivedere la natura giuridica del rapporto di lavoro degli operai dell'ex Corpo forestale dello Stato, ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto privato. Com'è possibile che lo Stato ancora non risolva tale questione? Vi sono inoltre le proposte che riguardano gli animali, formulate dalla deputata Sarli, che mi ha chiesto di depositarle a mio nome, visto che alla Camera il bilancio arriverà blindato (anche questa è prassi consolidata). Tali proposte prevedono la riduzione dell'aliquota IVA sul cibo per gli animali e sulle prestazioni veterinarie dal 22 al 10 per cento e di aumentare l'importo massimo delle spese veterinarie detraibili fino a 650 euro, in luogo degli attuali 550. Eppure, noi sappiamo - come ci dice anche il rapporto Assalco-Zoomark del 2021 - che sono circa 60 milioni gli animali da compagnia e non si può

creerà un effetto finanziario, in termini di casse dello Stato, pari a meno 393 milioni di euro fino al 2025 per la plastica e meno 462 milioni di euro fino al 2025 per la tassa sui prodotti dolciari, senza dimenticare ovviamente gli effetti negativi per l'ambiente, l'economia e la salute dei cittadini. Da che parte stanno lo Stato e la maggioranza? Dalla parte delle grandi imprese e dei più forti? È così, non c'è dubbio. due esempi per tutti, che hanno mobilitato in queste settimane lavoratori e cittadini, ma senza successo, perché il Governo ha deciso di stare dalla parte dei più forti e semplicemente ignorare le buone proposte, come quelle che abbiamo fatto noi. Mi riferisco, in

con il pagamento di una penale, quando invece bisognerebbe chiedere la restituzione dei contributi pubblici ricevuti dalle aziende. C'è poi il tema dell'autonomia differenziata: si rischia di allargare la differenza tra Nord e Sud. In piazza ieri c'erano molte persone, ma forse ancora poche, perché il Sud lo stiamo abbandonando. Qualche settimana fa la Corte costituzionale ha valutato negativamente il ritardo dello Stato nella definizione dei livelli essenziali essenziali delle prestazioni, (LEP) precisando che bisogna definirli con urgenza, anche in vista di un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Inoltre, la Corte dice che il ritardo delle definizioni dei LEP rappresenta un ostacolo non solo alla piena attuazione dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, ma anche al pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti sociali.

ci impone di controllare il Governo. Questo continuerò a fare, nonostante il Governo stia ribaltando i ruoli e, giorno dopo giorno, stia sottraendo spazi di democrazia al Parlamento. I cittadini devono sapere che è a rischio la loro rappresentanza.

non è possibile l'alterazione del rapporto tra Governo e Parlamento attraverso l'utilizzo della legge di bilancio per inserire alcune norme, in particolare riforme, che il Governo ritiene di dover adottare, senza il pericolo - sottolineo pericolo

Mi soffermo quindi su una questione specifica che rappresenta quello che sto dicendo. Gli emendamenti proposti dal Ministero della giustizia in materia di giudici onorari

Presidente, se lei va a vedere, era la prima volta che l'articolo 186 prevedeva una copertura di un provvedimento che non c'era. Abbiamo sempre visto provvedimenti mancanti di copertura. Questa volta avevamo una copertura per un provvedimento che ancora non c'era. Ne abbiamo discusso la settimana scorsa in Commissione e, su mia proposta, all'unanimità, Presidente, abbiamo rivolto un appello al Ministro della giustizia affinché non presentasse questi emendamenti,

di sbavature? Dobbiamo tener conto che, quando si parla di magistratura onoraria, ci sono due atteggiamenti, che sono

onorari attraverso il riferimento a una determinazione di stipendi che riguardano i dipendenti della pubblica amministrazione. Lei mi insegna che una è una determinazione di legge, mentre l'altra è un effetto della decisione contrattuale sugli stipendi dei pubblici dipendenti. Che cosa avverrà se quello stesso stipendio cui si fa riferimento nella norma viene aumentato in sede contrattuale? L'altro, che è determinato per legge, dovrebbe essere aumentato automaticamente? Non si capisce nulla. nulla. Io mi limito a questo, Presidente. Vorrei tanto che ci fosse la possibilità - e lo chiedo al Ministro della giustizia - di fare in gennaio una riflessione seria, perché nella vita bisogna pur capire che a volte la riflessione immediata può portare a correzioni utili. *(Applausi)*. Signor Presidente, rappresentante del Governo, svolgerò alcune rapide considerazioni sul disegno di legge di bilancio al nostro esame. In premessa, voglio anch'io associarmi ai ringraziamenti corali che sono stati rivolti a tutti i senatori commissari, che hanno lavorato incessantemente durante le scorse ore per portare in porto questo importante provvedimento. Mi sia consentito, consapevole che

Se qualcuno mi dovesse chiedere se sono soddisfatto di questo disegno di legge di bilancio, da senatore della Repubblica che rappresenta la Nazione e considerata la situazione di contingenza nella quale ci troviamo, ossia di perdurante emergenza sanitaria, economica e sociale, non potrei che rispondere affermativamente: sì, sono soddisfatto. Non potrebbe essere diversamente,

non posso che essere soddisfatto, se si considera anche l'importante investimento di 4 miliardi per contenere l'aumento delle bollette di luce e gas. Su questo però è doveroso aprire una parentesi. Così come è stato ribadito ieri da Matteo Salvini, questo è un importante provvedimento, che riguarda questo momento, questo istante, ma non è bastevole per affrontare il prossimo futuro. Non a caso, il nostro segretario federale ha

con una rateizzazione in dieci mesi, dall'altro lato dobbiamo considerare le numerosissime aziende e imprese che stanno andando in sofferenza. Da sindaco, posso anche esprimere felicitazioni per l'intervento che vi è stato in merito alla TOSAP, la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, nei confronti delle attività commerciali, dei ristoratori, dei bar e di tutti gli esercizi pubblici; sappiamo che anche questo tipo di intervento è un aiuto molto importante.

Vigili del fuoco siano equiparati a quelli di tutte le Forze dell'ordine. Un motivo per essere felici è anche l'importante stanziamento (30 milioni di euro) previsto per l'autismo: significa dare un concreto aiuto a famiglie che soffrono in silenzio e che fino a ieri soffrivano dimenticate. Sappiamo però benissimo che con l'ottimo lavoro del ministro Stefani questo non accadrà più. Siamo parimenti

parte attiva, proponendo subemendamenti che avrebbero migliorato ulteriormente il provvedimento. Passo a una considerazione riguardante l'ambito più territoriale. Ho sottoscritto un emendamento, a prima firma

Mi ricollego a quanto detto saggiamente ieri dal senatore Candiani. La legge di bilancio non può essere il ricettacolo delle mille sollecitazioni che giungono dal territorio, ma deve avere una visione ampia e considerare i settori nella visione dell'intera Nazione in maniera quanto più strutturale possibile e non parcellizzata.

la tagliola rispetto a determinati provvedimenti sia messa dalla burocrazia o da qualche Sottosegretaria che ritiene di fare la maestrina, invece che il rappresentante del Governo.

di buon Natale a tutte le italiane e a tutti gli italiani, senza asterischi, perché siano sempre fieri

per il 2022 ha un'importanza ancora maggiore, considerando il contesto sanitario, sociale ed economico in cui ci troviamo. La legge di bilancio in esame, che contiene misure per circa 37 miliardi, rappresenta un crocevia fondamentale per le sorti e il futuro dell'economia italiana, dopo quasi due anni di paura e di incertezza determinati da questa pandemia. Al nostro Paese oggi serve quindi una legge di bilancio coraggiosa, che sia espansiva, orientata alla crescita e tesa a contemplare tutte le diverse esigenze dei cittadini e delle imprese. Per il MoVimento 5 Stelle la legge di bilancio è un esercizio molto delicato e complesso, volto a mettere davanti il bene collettivo, anche rispetto agli interessi personali e al consenso politico, perché il MoVimento 5 Stelle non fa emendamenti a tornaconto elettorale o territoriali, ma si fa carico dei problemi della comunità che toccano tutti quanti in egual misura cercando di non creare cittadini di serie A e cittadini di serie B, in una logica che ci vede sempre soli in queste battaglie. Vorrei fare anche qualche esempio:

alle ore 5 di mattina siamo da soli a difendere questo provvedimento, cercando di portarlo a casa. Questo è il modo con cui stiamo lavorando. Lo facciamo per difendere tutti, senza nessun problema, perché abbiamo come unico faro il bene comune. comune. *(Applausi)*. Un altro esempio che mi viene in mente è che il MoVimento 5 Stelle è l'unica forza politica che difende chi si trova in povertà, anche solo momentaneamente per i motivi causati dal Covid, che hanno accentuato le difficoltà delle persone, che oggi non sono più sole,

L'abbiamo protetta anche dai cosiddetti Robin Hood dei poveri, che vogliono spostare i soldi del reddito di cittadinanza e li vogliono portare ad altri poveri. Ciò non ha senso: queste persone vanno aiutate e noi ci siamo, anche per i rincari delle bollette, che - tengo a ricordarlo - sono altissimi, perché sono frutto delle politiche sbagliate di questo Paese che si è continuato a legare alle fonti fossili. qualcuno qui in Aula sogna e parla del nucleare, lo sentiamo continuamente, tutti i giorni. A queste persone dico di farsi promotori di un *referendum,* di farsi dare i pieni poteri dai cittadini e di tornare qui a parlare di nucleare.

risorse preziose, che sosterranno una manifestazione sportiva molto importante dedicata ai giovani, seguita a livello internazionale, ma che può mostrare a tutto il mondo la bellezza e il fascino del nostro Paese. di una manifestazione dedicata allo sport giovanile, ai giovani, che per due anni hanno veramente combattuto con noi in questa pandemia. C'è una grandissima difficoltà ad organizzare questi eventi nazionali che portano ricchezza e danno

con la sua carovana colorata, toccherà tante Regioni del nostro Paese, da Nord a Sud ed è un'occasione per valorizzare il *made in Italy* attraverso uno sport che affascina i giovani che lo praticano. Ringrazio anche il ministro Di Maio per avermi supportato nella realizzazione di questo evento di questo emendamento, che sarà sicuramente un forte traino per l'economia di scala, che si crea quando tali eventi vengono realizzati. Ci sarebbero però tanti emendamenti di cui parlare, sui quali abbiamo lavorato. L'interesse collettivo sarà sempre il faro del MoVimento 5 Stelle, indipendentemente dal consenso elettorale. Non troveremo mai emendamenti su una piscina, su una strada, su un lungomare, su assunzioni di personale o su un campo sportivo, perché il nostro unico obiettivo è il bene comune. Dobbiamo ricordarlo sempre, perché noi rispondiamo a tutti i cittadini. Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, rappresentanti del Governo, dalla nascita di questo Governo siamo spesso stati accusati, come Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia, di fare inutilmente opposizione a un Esecutivo autorevole, nato con la finalità di traghettare l'Italia fuori dal guado in cui i precedenti Governi l'avevano portata. Tuttavia, è giusto sempre ricordare che è un bene che ci sia un'opposizione oggi in Aula, non solo per il Parlamento, ma anche per l'intero Paese, che può vantare un gruppo di rappresentanti che, con senso critico, ma costruttivo, sono a vigilare sull'operato di un Governo che non smette di non convincerci. Cari colleghi, dico ciò perché, come ha detto la nostra Presidente nazionale, Giorgia Meloni, oggi siamo in quest'Aula a fare un'opposizione seria, lucida e patriottica, che non si limita a votare a favore o contro ogni vostra proposta, ma che anzi desidera far sentire la nostra voce e le nostre argomentazioni. Nonostante i buoni propositi dei parlamentari di Fratelli d'Italia, tuttavia, ci troviamo a discutere di una prerogativa fondamentale del Parlamento, la legge di bilancio, con tempistiche molto, troppo troppo strette, senza una possibilità di manovra rilevante. Ciò è frutto di un atteggiamento preciso dell'Esecutivo nei confronti del potere legislativo, troppo spesso messo sotto scacco dal Governo mediante il voto di fiducia, nonostante all'opposizione ci siamo solo noi. L'indicazione di Palazzo Chigi sembra infatti quella di passare oltre le prerogative del Parlamento anche stravolgendo la democrazia parlamentare. però, abbiamo il compito, affidatoci dagli italiani e dalle italiane, di far sentire la nostra voce il più possibile. Come sottolineato ieri dalla senatrice Rauti, Fratelli d'Italia ha presentato 700 emendamenti, senza la pretesa che venissero tutti approvati. Come precisato dalla stessa collega, però, ci siamo dovuti scontrare contro un muro di gomma, che ha rifiutato qualsiasi proposta provenisse dai nostri banchi. Oggi siamo qui, signor Presidente, per votare una manovra che riteniamo non essere la migliore per noi italiani, quegli stessi italiani, non devo essere certo io a ricordarlo, che ancora oggi non hanno superato i danni atroci che abbiamo ereditato da una pandemia che ancora ci attanaglia. È un danno sociale, ma certo anche economico, molto rilevante, arginare - bisogna farlo - con una politica sociale ed economica mirata. Tra i più colpiti ci sono stati gli imprenditori, piccoli e grandi, di qualsivoglia settore. È triste annotare che questo Governo, troppo miope, non ha mai attuato un piano di aiuti funzionale come noi di Fratelli d'Italia chiediamo da tempo. Lo stesso Governo, invece, con questa manovra fiscale si è preoccupato di reperire una quantità enorme di denaro pubblico per finanziare nuovamente uno dei più fallimentari interventi di politica economica della storia repubblicana, ossia il reddito di cittadinanza, uno strumento di sussidio inutile, anzi dannoso, che si è dimostrato inefficace in molteplici occasioni. Anche su questo tema siamo spesso stati attaccati, ma la verità è che il reddito di cittadinanza, come più volte detto in quest'Aula, serve solamente a mantenere persone che non sono inabili al lavoro per sfortuna o contingenza. Questo strumento serve solo a coloro che non vogliono produrre ricchezza per la collettività, lasciando nuovamente in un angolo quelli che un impiego realmente lo cercano e ne hanno la necessità,

giunti in Italia una sola volta, se ne sono andati con i soldi destinati ai cittadini italiani. Ovviamente siamo consapevoli e riconosciamo che vi sia una categoria di cittadini, di uomini e donne, che va aiutata, tutelata e inserita in modo graduale e controllato nel mondo del lavoro ed è ancora più sconfortante annoverare che nemmeno con un tale esborso di soldi pubblici si sia trovato un impiego a dette persone. Infatti, anche per i disabili - dati alla mano - il reddito è stato fallimentare. Riteniamo che il denaro pubblico debba essere investito sulle aziende, ossia su chi crea ricchezza, cosicché ne possano poi fruire i cittadini sotto forma di salari e stipendi. Invece, per l'evidente colpa di uno schieramento politico e della propria cecità, lo Stato non riesce a utilizzare al meglio i propri fondi. Questo denaro potrebbe essere impiegato in modo migliore, ad esempio nel credito da erogare alle imprese italiane, le quali non solo sono in un momento di sofferenza economica, ma sono anche abbandonate dallo Stato e dalla politica. È nostro dovere, pertanto, trovare una soluzione per cercare almeno di arginare la grave perdita dal punto di vista economico, anche perché in un periodo di crisi economica non solo, com'è ovvio, non gioverebbe alla Nazione, ma, considerando il contesto - ora storico, ora geopolitico - provocherebbe un vantaggio enorme verso la concorrenza di altri Stati economicamente aggressivi come la Cina. Purtroppo oggi siamo invece in quest'Aula a esaminare con vergognoso ritardo una manovra di bilancio lontana dalle esigenze del tessuto produttivo italiano e vicina a quello passivo. Noi, al contrario, siamo sempre dalla parte di chi sceglie di fare impresa e non è solo uno *slogan*, perché è pacifico che le aziende sono il motore del Paese e senza questo motore il Paese non si muove. A noi piace tuttavia parlare di cose concrete e da imprenditore, nonché da cittadino che ha a cuore le sorti delle nostre aziende, eccellenze in molteplici settori, tengo a sottolineare che il sostegno pubblico alle imprese, che per inciso doveva essere assicurato anche mediante i finanziamenti bancari interamente garantiti dallo Stato, ai sensi della normativa di emergenza, è risultato lacunoso e non in grado di supportare tutte le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria. È superfluo e assolutamente pretestuoso voler spiegare in quest'Aula l'importanza del provvedimento e, soprattutto, la portata del danno cagionato dalla sua mancata messa in opera. La conseguenza è stata la chiusura di moltissime imprese e quindi cittadini senza impiego e senza mezzi di sostegno per provvedere ai propri bisogni e a quelli delle famiglie. Se avere centinaia di migliaia di cittadini che faticano ad arrivare a fine mese e a portare il pane a tavola non è un problema per questo Esecutivo, bisogna altresì annoverare che le aziende che hanno chiuso i battenti sono in larga parte operanti in settori strategicamente fondamentali per l'Italia, quali il turismo, il commercio e la ristorazione. A proposito della ristorazione è opportuno e doveroso citare il pessimo trattamento riservato ai ristoratori nell'arco della pandemia, i quali, nonostante abbiano di euro per ottemperare alle norme vigenti e porre il proprio locale in sicurezza, si sono trovati più volte a dover abbassare la saracinesca. Per questo vi è la necessità e l'estrema urgenza di porre in atto un procedimento in favore delle tante e troppe attività imprenditoriali in sofferenza, anche considerando - non è un fatto secondario - l'enorme gettito fiscale che le aziende versano nelle casse dello Stato, nonché gli spropositati aumenti dei costi per l'energia, che hanno minato la stabilità di aziende perfettamente in ordine e funzionanti nell'anno corrente e che sono una minaccia al mantenimento in vita del nostro tessuto economico nel 2022.

di poter vivere una vita in condizioni adeguate come la politica deve saper garantire.

possono celebrarlo. Chissà se le nuove generazioni riusciranno a festeggiarlo, visto l'attacco progressista

Cercherò di arrivare subito al nocciolo della questione, dato che il tema oggetto dell'emendamento bocciato da questa maggioranza riguardante le patenti è stato già affrontato.

costi 2.500 euro e nel Regno Unito 250. Ne abbiamo discusso in Commissione; abbiamo provato a sollecitare il Sottosegretario, il Ministro e i commissari.

a fronte di quanto si guadagna in altre nazioni europee. Il costo della formazione chiaramente penalizza oltremodo i lavoratori italiani. italiani. Andava garantito, quindi, un supporto economico proprio per avviarli al mondo del lavoro. Si parla dell'introduzione dei giovani della grande questione lavorativa e poi lo Stato si gira dall'altra parte. Continueremo a ripeterlo: secondo noi, in Italia costa troppo prendere una patente di guida per

Il Governo pensa di aver risolto la questione con il *bonus* patente. Abbiamo chiesto di allargare la platea di coloro che potevano usufruire di questa possibilità anche ad altre categorie di autisti e ad altre tipologie di autotrasportatori, ma l'emendamento è stato clamorosamente pertanto che sono qui ad esprimere, a nome di tutto il Gruppo Fratelli d'Italia, il nostro disappunto e la nostra delusione, una critica purtroppo dura,

migliaia di posti di lavoro e consentito a migliaia di giovani di essere in linea con quanto accade nel resto d'Europa. resto d'Europa. Rispetto a questa drammatica carenza di autisti, ci siamo sentiti rispondere ancora una volta no.

Non è più accettabile tutto questo; l'abbiamo denunciato, ci siamo battuti, abbiamo provato, anche con le armi della diplomazia, a far riflettere questo Governo. Il risultato è quello siete rimasti sordi a questa esigenza della Nazione (non è un'esigenza nostra). Sono qui appunto - e ho concluso - a rappresentare tutto il mio sdegno e la mia delusione.

di quel Governo e anche nell'ambito delle stesse maggioranze ci fu chi ammise che non era questo il sistema. Bene, qui abbiamo superato di gran lunga tutti i peggiori *record*, anche degli ultimi anni. Ricordo che, fino a non molti anni fa, solo il fatto di porre la fiducia sulla legge finanziaria era visto come una cosa estremamente discutibile, come un atto criticabile, perché comprime la possibilità del Parlamento di esprimersi.

spesso non hai modo di difenderti. Bene, lo Stato, nel momento più importante dell'anno dal punto di vista finanziario, ma anche dell'intera linea politica del Governo,

Nella sostanza, il disegno di legge di bilancio denuncia tutti i problemi di una maggioranza estremamente variegata e diversa come linee, come esigenze,

ci siano dei voti, dei sì e dei no, e possibilmente, quando il Governo dice no, dovrebbe anche spiegarlo. Fino a pochi anni fa i relatori non facevano solo i lettori

in altri casi risiede in potentati che non hanno nulla a che fare con il consenso popolare, ma a volte godono di un forte potere che esercitano in vari modi. Per esempio, il Ministero dell'economia e delle finanze, con i suoi autorevoli rappresentanti nella Commissione, ha dovuto dire una serie di no - questo è ovvio - a tante proposte che, come è normale per un disegno di legge di bilancio, chiedevano l'impiego di denaro.

anni di interrogazioni in merito, abbiamo finalmente potuto sentire una rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze parlare dell'affare Autostrade Aspi, dove il Governo, senza darlo a vedere, ma soprattutto senza informare rigorosamente il Parlamento, nonostante le numerose interrogazioni di esponenti sia della maggioranza sia dell'opposizione,

Hanno fatto crollare il Ponte Morandi o diciamo che sotto la loro gestione è crollato il ponte Morandi; la magistratura ha preso provvedimenti molto chiari, l'avvocatura dello Stato ha detto che c'erano gli estremi per la risoluzione per inadempimento da parte del concessionario.

Da questo deriva la seconda mossa del Governo, che sta rinunciando al diritto di recesso previsto dalla convenzione approvata in Parlamento nel 2007, che concede a ciascuna delle parti, in particolare al concessionario Stato, proprietario delle infrastrutture, ivi comprese le autostrade gestite dai concessionari privati, la possibilità di recedere in qualunque momento dal contratto, pagando determinate somme su determinati parametri che sarebbero in questo caso 13,8 miliardi. Ebbene, il Governo sta facendo un affare, guidato da Cassa depositi e prestiti, per dare ad Atlantia, ossia i signori Benetton con gli altri rispettabilissimi azionisti di Atlantia, la bellezza di 7,5 miliardi in più, come minimo. Questo supponendo che i tribunali diano torto dalla A alla Z al Governo, dicendo quanto hanno fatto bene i Benetton, come hanno fatto bene la manutenzione e che il ponte Morandi è crollato chissà perché. Pertanto, con che faccia il il Governo può dire di no alla proposta di rialzare le pensioni di invalidità, che magari costa qualche centinaio di milioni? Può dire di no a tagliare le tasse alle aziende che assumono e alla nostra proposta "più assumi meno paghi", che costerebbe forse qualche centinaio di milioni, quando poi si trovano, senza dire nulla al Parlamento, 7,5 miliardi da regalare a chi

stesse problematiche si risponda nella stessa maniera da parte del Governo.

una prosecuzione del regime di ammortizzatori sociali e comunque di sostegno per il 2022 e per il 2023. Alitalia, una società privata e non pubblica, anche se poi tra pubblico e privato c'è una commistione di cui non riusciamo a capire l'esatta portata, ossia se catalogarla come pubblica o come privata. L'altra società è Air Italy: cessa l'interesse della società, che intenderebbe non proseguire con l'attività, per eventuali malintesi o cessazione di interesse tra Qatar e il consorzio Costa Smeralda consorzio Costa Smeralda (ovvero Aga Khan). Ebbene, per questi lavoratori non si trova alcuna forma di sostegno, neanche forse per arrivare a fine anno e niente per il 2022. Si tratta di un problema di giustizia

oltre 1.300 persone - circa 1.300 famiglie - che rimarrebbero senza alcun sostegno fino a fine anno e per l'anno a venire. Dico questo veramente mi spinge un sentimento di ricerca di giustizia: non è pensabile che a problemi identici ci siano soluzioni diverse. Non parlo e non ho parlato di ciò che va bene della manovra e di ciò che va meno bene. Parlo invece di un problema di giustizia, e lo chiedo a nome dei

Di fatto, abbiamo una Camera che si occupa del provvedimento in Commissione (non in Aula, diciamocelo francamente) e un'altra Camera che, a fasi alterne, di anno in anno prende atto e, attraverso la fiducia, vota soltanto sì o no al provvedimento. È un atteggiamento inaccettabile, è qualcosa che deve essere modificato, perché altrimenti si sta verificando

che esiste di fatto, così come di fatto esiste soltanto l'attività legislativa di una Camera.

dal punto di vista di chi siede in Parlamento sia problematico portare il proprio apporto e le proprie idee per migliorare certi provvedimenti. Non è quanto dovrebbe accadere. Non vorrei arrivare al punto di dire ciò che disse qualche anno fa un nostro collega, che ho avuto l'onore di conoscere in quest'Aula e che ora non c'è più, ma è stato anche Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga:

un po' scherzava, un po' diceva la verità. Di fatto, noi non abbiamo la possibilità di conoscere pienamente quanto andiamo a votare; non lo sapete neanche voi, colleghi della maggioranza, che voterete a favore del provvedimento. Noi almeno voteremo contro e già con questo

Arriviamo a questo perché ci sono veti incrociati all'interno della maggioranza, mancette che vengono date a questo e a quell'altro e continue diatribe all'interno della maggioranza, che non si mette d'accordo. Noi però come Fratelli d'Italia e come opposizione, abbiamo portato

L'attenzione nei loro confronti deve infatti essere primaria nel nostro Paese, perché la sicurezza non è soltanto un argomento di cui si parla in campagna elettorale parla in campagna elettorale per dire che siamo tutti per la sicurezza; ci mancherebbe che qualcuno dicesse poi che è per l'insicurezza o per la delinquenza. Di fatto però quando il Parlamento, attraverso la manovra di bilancio, non aiuta

è un detenuto come gli altri, perché passa tantissimi anni in condizioni non facili, in cui è difficile stare a contatto con le emergenze sociali che si pongono in quell'ambito. In tutto questo sarebbe stato importante da parte del Governo stanziare più soldi possibili per le assunzioni. Anche per quanto riguarda la Polizia penitenziaria dei ragazzi che hanno fatto i concorsi sia per quanto riguarda il personale che proviene dal mondo delle Forze armate sia per quanto riguarda persone che hanno fatto concorsi civili e sono in attesa delle assunzioni che invece non vengono fatte. Voglio sperare che

sicurezza non è un argomento da trattare solo in campagna elettorale. Noi crediamo nella sicurezza sempre. Non ci si può scandalizzare quando succede il fatto grave o quando il poliziotto viene aggredito o quando qualcuno fa qualcosa per strada e non viene adeguatamente fermato; il Parlamento deve intervenire nei fatti, garantendo la sicurezza ai cittadini e dando la possibilità alle Forze dell'ordine di operare al meglio. *(Applausi)*. Signor Presidente, non farò alcuna considerazione di metodo. Mi asterrò dal commentare gli aspetti sui quali molti i colleghi sono intervenuti sull'*iter* parlamentare, anche perché rischierebbero di essere considerazioni troppo ingenerose e penso che la fase delicata che il Paese sta attraversando, sia dal punto di vista sociale, nel contrasto alla pandemia, sia sul fronte economico, non lasci a nessuno di noi lo spazio per la consenta tuttavia di dire, Presidente, che in questo passaggio cruciale la manovra di bilancio, a nostro giudizio, poteva e doveva essere più coraggiosa e più coerente. Lo dico da sostenitore di questo disegno di legge di bilancio e da membro della maggioranza. Poteva essere più coraggiosa e più coerente a partire proprio dalla

trova un evidente consenso tra i cittadini. Ma c'è un'urgenza, anzi un'emergenza in questo Paese. In politica, quando ci sono le emergenze, queste diventano priorità priorità dell'azione del Governo e del Parlamento in primissima battuta. L'emergenza di questo Paese si chiama lavoro giovanile: non c'è altra questione, dal punto di vista della riduzione delle tasse, che venga prima del ridurre una disparità inaccettabile, come ha ricordato recentemente pubblicamente Carlo Calenda, riprendendo i dati dell'Istat, che voglio ricordare a quest'Assemblea come punto di partenza. Il reddito medio annuo degli italiani è di 21.965 euro; il reddito medio degli *under* 30 è di 15.128 euro; il reddito medio degli *under* 25 è di 9.935 euro. Un giovane che lavora in Italia guadagna meno della metà del reddito medio. Ebbene, più coraggio e più coerenza avrebbero voluto dire almeno discutere l'emendamento che abbiamo presentato come Misto-+Europa-Azione. Signor Presidente, se 5,5 di quegli 8 miliardi destinati alla riduzione dell'Irpef fossero andati

soffermo su questo aspetto, perché non possiamo continuare con la retorica della questione giovanile, di cui riempiamo gli appuntamenti di partito, di ogni partito, e poi, quando è ora, avendo la possibilità di mettere in campo un provvedimento concreto, non farlo. Continuare con questo approccio sulla modifica delle tasse, dell'Irpef e dell'imposizione in generale, limando un po' scaglioni e aliquote, non fa altro che rafforzare quella odiosa ingiustizia che don Milani, nelle lettere alla professoressa, definisce le «parti uguali tra disuguali»: i disuguali oggi sono una generazione che ha un accesso al reddito semplicemente insopportabile. Presidente, mi consenta una considerazione velocissima sul tema della scuola. Il Governo ha fatto uno sforzo importante in questa manovra di bilancio, prevedendo uno stanziamento tra i più significativi degli ultimi anni

anche quello del raggiungimento di obiettivi importanti come il contrasto all'abbandono e alla dispersione scolastica. A questi aspetti nulla è legato in termini di riconoscimento economico. In Italia nel 2020 543.000 ragazzi hanno abbandonato gli studi. Sono percentuali drammatiche, che ci collocano al quarto posto, in termini negativi, in Europa. Dico questo perché sui temi della formazione, dell'insegnamento e dell'acquisizione delle competenze quest'Assemblea avrà un ruolo centrale. Penso alle prossime settimane, quando discuteremo la riforma e le modifiche che arrivano dalla Camera dei deputati. Voglio sperare che non ci sarà un arretramento su un livello strategico di preparazione dei nostri giovani rispetto a quanto fatto dalla Camera

credo che il senso profondo dell'azione politica si manifesti in due forme: guidare la Nazione verso una certa idea di futuro, sviluppo e benessere e sostenere chi non riesce a reggere il passo verso la meta indicata. È inutile negare che in questa fase eccezionale, nel pieno della crisi di sistema che stiamo vivendo, il primo compito è assolto in forma quasi esclusiva dal presidente del Consiglio Mario Draghi e dal suo Governo. Al Parlamento non resta - e non è poco - che assolvere, nei margini spesso ristretti che il Governo lascia, il secondo compito. Ciascuno di noi in quest'Aula per sensibilità personale, orientamento politico e provenienza territoriale

Il primo è cercare di sostenere fattivamente e concretamente i bisogni dei cittadini marchigiani e delle altre tre Regioni sconvolte dal terremoto del 2016, sapendo che, a causa di una carenza del sistema pubblico nel suo complesso, i loro bisogni non sono stati ancora soddisfatti. Il secondo riguarda lo stato dell'editoria, che è il mondo da cui provengo e non solo per questo ritengo doveroso occuparmene. Altri colleghi hanno parlato e parleranno delle vicende legate al terremoto, quindi concentrerò il mio breve intervento sul tema dell'editoria. Comincio col rammaricarmi perché diversi emendamenti che ho presentato non sono stati non hanno avuto il via libera del Ministero dell'economia; in particolar modo, uno tra i segnalati puntava alla forfettizzazione delle copie rese. Sarebbe stato un provvedimento utile

distributori, stampatori, produttori di carta, edicolanti e via elencando. Non mi nascondo e non mi illudo, perché, se anche fossero stati accettati tutti gli emendamenti che ho presentato, non per questo la situazione del comparto sarebbe cambiata in maniera radicale.

ma soprattutto oltre l'80 per cento dei ricavi da pubblicità. A questo stato di fatto si aggiunge che i costi di produzione stanno vertiginosamente crescendo: tanto per dare un unico elemento il costo della cellulosa è aumentato del 70 per cento. Stiamo parlando di una filiera che dà lavoro complessivamente a 90.000 persone.

della nostra democrazia intervenendo con risorse pubbliche. Proteggere l'editoria vuol dire proteggere e rafforzare il diritto dei cittadini di essere debitamente informati, rafforzare e dare loro degli strumenti per per orientarsi in un mondo che è quanto mai scombussolato, ha perso la bussola (si sono perse le gerarchie delle notizie, si è perso il senso della realtà) e per consentire loro di esercitare con cognizione di causa il proprio diritto-dovere di voto. Conoscere per deliberare diceva Luigi Einaudi e naturalmente diceva la verità. molto popolare soprattutto tra i ranghi di quel MoVimento 5 Stelle dove tutt'oggi c'è chi ha inteso e tuttora intende far morire per fame, affamare letteralmente editori e giornalisti, evidentemente volendo servire gli interessi dei giganti del *web.* Ebbene, Stiglitz diceva che l'informazione è un bene pubblico e in quanto bene pubblico ha bisogno di sostegno pubblico. Non è un vezzo, non è un capriccio, non è retorica; è quanto concretamente fanno tutti i Paesi civilizzati del mondo. Una ricerca di dieci anni fa dell'università di Oxford diceva che l'Italia è l'ultimo Paese tra quelli che sostengono attivamente la propria editoria nazionale; i dati più recenti della Banca mondiale confermano, purtroppo, questa tendenza. Il Paese che più si spende e spende per l'editoria è la Danimarca con 9,59 euro per abitante, in coda alla classifica c'è l'Italia con 1,49 euro: quasi 10 euro per cittadino

e questo potrebbe anche andar bene, perché il mondo cambia, la rivoluzione digitale ha cambiato il mondo, cambiano le abitudini, alcune professioni scompaiono, altre nascono, cambia anche il modo di informarsi dei cittadini, se non fosse che quelle fonti sono prevalentemente "avvelenate". Vi fornisco alcuni elementi di fatto che forse, coniugati e letti in sequenza logica, fanno un ragionamento: (MIT) di Boston afferma che sui *social* in generale e su Twitter in particolare le notizie false si diffondono sei volte più velocemente delle notizie vere.

contestualizzarli, capirne il senso e comprenderne la portata. Eppure, mai come oggi l'opinione pubblica ritiene di essere iperinformata. I rapporti OCSE Pisa ci dicono che i nostri figli, i nostri nipoti, quando si informano guardando un sito *web* non riescono a distinguere tra un contenuto pubblicitario e un'informazione, una notizia. Non distinguono tra pubblicità e notizia, tra la parte teoricamente giornalistica e quella evidentemente pubblicitaria. Le ricerche americane dicono che la lettura su carta s'imprime enormemente di più nella memoria e stimola enormemente di più il pensiero rispetto alla lettura su dispositivo digitale, ancor più naturalmente rispetto alla fruizione dei medesimi concetti attraverso Se abbiamo a cuore, non la quantità delle informazioni, ma la qualità dell'informazione, questi dati dicono che il digitale, evidentemente, non è un degno sostituto della carta stampata e che i *social* non sono un degno un degno sostituto dei giornali. Ora, conosco la serietà e la dedizione del sottosegretario all'editoria Giuseppe Moles e ho apprezzato molto il fatto che sia stato inserito, nelle pieghe di questa legge di bilancio, un fondo straordinario per l'editoria. Non ho dubbi sul fatto che il Governo recepirà nel migliore dei modi il piano cui sta lavorando l'intera filiera dell'informazione e che lo saprà inserire adeguatamente nel PNRR, per consentire a questo comparto di adeguarsi al cambiamento e alla transizione digitale. saranno poi i giornalisti e gli editori a doversi dimostrare all'altezza di questo compito, un compito che, mai come oggi, in un'epoca di grande caos, di grande confusione, che ha perso ogni principio ordinatore, non è esagerato definire storico. Un compito del genere va assolto con senso dell'onore personale e soprattutto con senso di responsabilità nazionale. In questi giorni, soprattutto alla luce di quanto detto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, due giorni fa, sul rapporto malato tra

non deprimere l'umore dei combattenti al fronte e dei concittadini in Patria. Vi lascio con questa riflessione. Non aggiungo nulla. Una riflessione a partire da questo punto sarebbe opportuna, non certo in un'Assemblea parlamentare ma tra i ranghi della categoria cui appartenevo.

colleghi, signori Sottosegretari, innanzitutto desidero ringraziare i colleghi della 5a Commissione per l'impegno di queste ultime settimane, un lavoro stancante e senza sosta. Ma se ora vi chiedessi quali sono le cose più preziose della vostra vita, credo di poter ipotizzare, senza paura di essere smentita: la famiglia, i nostri cari e la salute. Nei momenti in cui la salute viene meno, vogliamo soprattutto due cose: innanzitutto essere curati e curati bene e poi avere accanto a noi le persone che amiamo, i nostri cari. Quindi, come istituzioni abbiamo il dovere di garantire l'accesso alle cure e la gratuità delle stesse.

Dicevo che, come istituzioni, abbiamo il dovere di garantire l'accesso alle cure e la gratuità delle stesse a tutti i cittadini, controllando la spesa e l'impiego delle risorse. Ogni singolo centesimo, infatti, deve essere impiegato in modo corretto e questo possiamo farlo solo con un sistema di tracciamento della spesa che garantisca la massima efficacia e responsabilizzazione. Siete davvero convinti che questo sia avvenuto negli ultimi due anni? Se - da un lato - è aumentato il fondo sanitario forse - dall'altro - vanno incrementati i controlli della spesa e degli impieghi. Tra l'altro - non so se ve ne siete accorti - ma, nonostante l'aumento del fondo, le liste delle visite specialistiche si allungano, gli *screening* non vengono fatti e gli interventi rinviati, con un danno inimmaginabile per chi si trova in condizioni di bisogno. In questa legge di bilancio, per fortuna, sono state approvate delle proposte emendative presentate in modo trasversale da tutte le forze politiche in tema di sanità: voglio ricordare la proposta sulle malattie retiniche, quella sul registro per la sclerosi multipla e molte altre che hanno visto tutte le forze partitiche lavorare nella stessa infatti solo il Covid, ma ci sono tutte le altre patologie - non solo quelle oncologiche - che non si fermano e non è più possibile procrastinare degli interventi di sistema. Tuttavia, si poteva e si doveva fare di più. Servono risposte vere e urgenti. le persone che saranno curate in ritardo vedranno compromessa la loro qualità di vita e, se non cambierà l'approccio, i costi sociali ed economici saranno inaccettabili e graveranno tutti sulle future generazioni. Su una manovra da 30 miliardi al Parlamento è stata data la possibilità di incidere per circa 600 milioni, briciole sostanzialmente. Poi c'è stata la tagliola degli emendamenti segnalati, per cui quelli troppo onerosi vanno Urge dunque una seria riflessione, perché in una Repubblica parlamentare le istanze raccolte dai parlamentari sono quelle degli italiani, mentre negli ultimi anni siamo stati trattati come acefali, chiamati a ratificare decisioni già prese. Parlando di salute, signor Presidente, voglio soffermarmi su un emendamento che non è stato considerato, né nel decreto fiscale, né nella legge di bilancio, non sicuramente per demerito dei colleghi, ma perché comporta Ad oggi chi è immobilizzato a letto e ha necessità di personale non specialistico per i propri bisogni quotidiani, per bere o mangiare, non può portare in detrazione le relative somme

ma devo dire che il deserto dei Tartari forse è più popolato in termini di risposte rispetto a quelle che abbiamo avuto in questa legge di bilancio. È un emendamento che costa, certamente. Ma ditemi, se voi foste bloccati a letto dal collo in giù, che cosa vi aspettereste dalle istituzioni?

È stato invece approvato un emendamento da 5 milioni per la sterilizzazione dei cinghiali. Siamo davvero sicuri che la sterilizzazione di questi mammiferi

Altro tema è il reddito di cittadinanza, che è stato finanziato in questa legge di bilancio per 8,4 miliardi complessivi, nonostante le continue truffe giornaliere che riempiono le cronache. Sicuramente è importante aiutare chi soffre, chi è più sfortunato, chi sta attraversando un momento difficile, ma perché non utilizzare quelle risorse per le aziende in crisi e per creare posti di lavoro? sappiamo tutti che trovare un lavoro nel Mezzogiorno è difficile, ma il presidente Draghi in questa Aula

all'inclusione sociale. Inoltre, al Mezzogiorno andranno altri 60 miliardi dei fondi strutturali e per lo sviluppo. È una valanga di soldi. Noi come Lega vigileremo affinché tutti vengano utilizzati in modo corretto, perché non si può solo chiedere; è fondamentale utilizzarli bene, perché coloro che dovranno restituirli sono i nostri figli. siamo un Governo di unità nazionale. La legge di bilancio rispecchia le diverse sensibilità e come Lega abbiamo avuto un occhio di riguardo per le bollette, l'Irpef, l'IRAP, il superbonus, l'APE sociale, la disabilità, cioè famiglie, partite IVA e aziende, ma per altri interventi siamo davvero lontanissimi. Lo sappiamo che rappresentiamo una spina nel fianco del Parlamento. I nostri emendamenti hanno sempre una strada in salita. Gli uffici ministeriali hanno difficoltà a fare le nostre ma pensate veramente con questi mezzi di fare un dispetto alla Lega? Lo fate ai cittadini italiani e noi, che da sempre li mettiamo al primo posto, continueremo a proporre i temi vicini alle esigenze della gente e decisamente lontani dagli interessi dei palazzi dove tanti

Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, le caratteristiche geografiche, geologiche e antropiche del nostro Paese lo rendono particolarmente vulnerabile ai rischi naturali, all'inquinamento delle matrici ambientali, al depauperamento del paesaggio e della biodiversità. Le sole alluvioni ogni anno mietono mediamente una ventina di sacre vite e generano danni per circa due miliardi e mezzo di euro. All'atavico elevato rischio idrogeologico si aggiungono gli effetti del cambiamento climatico, che rende più intensi e frequenti gli eventi meteo estremi. I terremoti poi sono come una spada di Damocle che statisticamente ogni quattro o cinque anni si abbattono violentemente sui nostri tanti territori a elevata pericolosità sismica e vulnerabilità. Solo negli ultimi tre grandi terremoti (L'Aquila, Emilia e Centro Italia) hanno cessato di battere 628 cuori e ci sono stati 44 miliardi di danni. 620.808 frane, valanghe, erosione costiera, emissioni di gas pericolosi, 158.000 ettari di bosco andati in fumo nell'ultima torrida estate, inquinamento delle acque e dell'aria. Come si può pensare di conciliare un qualsiasi sviluppo socio-economico sostenibile o transizione ecologica con tutti questi rischi che minano la sicurezza del territorio? È sacrosanto dovere della politica invertire rotte di collisione catastrofiche e dirigere la Nazione verso i sereni orizzonti di uno sviluppo ecosostenibile ed eticamente compatibile. Una sicura occasione per farlo è la legge di bilancio finanziando monitoraggio, previsione, riduzione, mitigazione e prevenzione dei rischi naturali e antropici, investimenti a grande moltiplicatore, sapendo che prevenire - per esempio - il rischio idrogeologico costa un quarto dei relativi danni e addirittura un decimo nel caso del rischio sismico. Badate bene: il fondamento della prevenzione è la conoscenza. Su questo concetto tornerò alla fine dell'intervento. Questa legge di bilancio interviene in modo importante sulla spesa primaria per la protezione dell'ambiente e per l'uso e la gestione delle risorse naturali. Sono previsti circa 9 miliardi e mezzo di euro per il 2022, il 59 per cento in più di quanto stanziato nel 2021. La maggior parte delle risorse iniziali interessa la protezione dell'area e del clima, ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente, protezione e risanamento del suolo e delle acque, protezione della biodiversità e del paesaggio. Per la riduzione delle emissioni climalteranti si istituisce un fondo per la mobilità sostenibile di circa 2 miliardi di euro fino al 2034; si istituisce il fondo per il clima di 840 milioni di euro per ciascun anno dal 2022 al 2026.

L'articolo 139 finanzia la spesa complessiva di 35 miliardi di euro fino al 2036 per interventi relativi alla manutenzione straordinaria e all'adattamento ai cambiamenti climatici della viabilità stradale regionale, provinciale e comunale. Vengono incrementati i contributi degli enti locali per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa a interventi di messa in sicurezza del territorio. Questo è un *vulnus* in Italia. La Corte dei conti ce lo ricorda ogni volta; nella relazione del 25 ottobre scorso è ben messo in evidenza che una mancanza è proprio la mancata progettazione di questi interventi. Si prevede un fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e dei reticoli idrografici. Viene rifinanziato con 200 milioni di euro, dal 2024 al 2029, il fondo per la prevenzione strutturale del rischio sismico e per studi di microzonazione sismica. La gran parte degli interventi per la tutela del territorio richiede un'approfondita conoscenza di base, che la moderna cartografia geologica al 50.000 può ben fornire. Ma tale cartografia è monca per colpa di un assurdo blocco di vent'anni dei relativi finanziamenti, mentre tutta l'Europa correva e oggi quasi tutte le nazioni non solo l'hanno completata, ma sono già agli aggiornamenti (al secondo, quarto o settimo aggiornamento). Ripartita grazie alle leggi di bilancio 2020 e 2021, ha ripreso grande vigore; ci aspettavamo che anche in questa legge di bilancio ci potesse essere la dovuta attenzione per rinforzare gli investimenti e renderli strutturali fino al completamento. Peccato che il Governo non abbia colto l'utilità universalmente riconosciuta di tale strumento di conoscenza basilare e non abbia provveduto a un adeguato finanziamento. Con una metafora clinica, potremmo dire che adagiamo un paziente con fratture multiple sul letto operatorio senza radiografie. Sì, la carta geologica ci fa operare consapevolmente e velocemente, ci fa risparmiare e salva la vita. Concludo: al mio personale dispiacere per tale mancanza governativa si contrappone la soddisfazione che il MoVimento 5 Stelle, unico e solo *(Applausi)*, sia stato sensibile, proponendo un emendamento che impegna 6 milioni di euro a tale scopo. Ciò evidenzia in modo inconfutabile quanto il MoVimento 5 Stelle sia attento ai reali bisogni della gente, alla sicurezza del territorio, alla prevenzione dei rischi naturali e alla vita. Sarebbe auspicabile che la necessità della conoscenza di base per qualsivoglia prevenzione diventi patrimonio condiviso di tutti. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza il calendario dei lavori fino all'11 gennaio. Nella giornata di oggi proseguirà, fino alla sua conclusione, la discussione generale sul disegno di legge di bilancio; seguiranno le repliche dei relatori e del Governo. Nella giornata di domani, a partire dalle ore 9,30, sarà discusso, anche ove non concluso in Commissione, il decreto-legge in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, già approvato dalla Camera dei deputati. Per la discussione generale sono state ripartite due ore e venti minuti in base a specifiche richieste dei Gruppi. Gli emendamenti per l'Assemblea dovranno essere presentati entro le ore 16 di oggi. L'ordine del giorno della seduta di domani prevede inoltre il seguito della discussione del disegno di legge di bilancio che proseguirà anche venerdì 24 dicembre. L'orario di tale seduta potrà essere anticipato in relazione all'andamento dei lavori. Il calendario potrà essere integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126*-bis*, comma 2-*bis* del Regolamento, sulla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. L'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 11 gennaio, alle ore 16,30, con la discussione delle ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri. Per le sedute successive la Conferenza dei Capigruppo sarà convocata nella stessa giornata di martedì 11 gennaio

che temo, però, cadrà nel vuoto, rispetto al fatto che non è consentito all'opposizione - vorrei dire all'intero Parlamento, ma parlo per la parte di questo Parlamento che rappresento

del Consiglio Draghi - è l'argomento fondamentale dello sviluppo dell'Italia nei prossimi anni. Ebbene, al Senato della Repubblica, all'unica forza di opposizione è chiesto di approvarlo a scatola chiusa, a scatola chiusa, senza leggerlo, senza sapere cosa c'è scritto, senza tentare perlomeno di emendarlo per la parte in cui è emendabile, di migliorarlo. Noi siamo chiamati esattamente a fare questo, presidente Calderoli e colleghi, ma pare che a nessuno più interessi pare che a nessuno più interessi cosa svolge il Senato, a cosa serve il Senato della Repubblica. Lo chiedo a voi: a cosa serve il ruolo che svolgiamo? Perché siamo qui, Presidente? Perché siamo qui, colleghi, se poi oggi, assumendovi una grave responsabilità, imponete al Senato di approvare un Piano dal cui funzionamento dipende il futuro dell'Italia senza avere la possibilità nemmeno di leggerlo? *(Applausi)*. È una cosa accettabile? È questa la democrazia dei migliori, Presidente? Provo vergogna per il fatto di non poter rispondere ai miei elettori su quello che oggi voi delibererete in 5a Commissione. Ricordo a lei, Presidente, che per vostra volontà, per vostro ritardo, per vostra incapacità, il disegno di legge di bilancio è stato approvato ieri alle ore 16 in Commissione bilancio dopo ventiquattr'ore di dibattito, e non per l'ostruzionismo di Fratelli d'Italia, che si è dimostrata ancora una volta opposizione irresponsabile, ma per vostra incapacità, per i vostri ritardi, per l'ostruzionismo che la maggioranza ha fatto alla maggioranza stessa. Avremmo potuto tenervi inchiodati per giorni in quella Commissione semplicemente chiedendo di votare tutti gli emendamenti, compresi i centinaia e migliaia di vostri emendamenti alla manovra, invece abbiamo deciso, per senso di responsabilità, perché ci teniamo a questa Repubblica e ci teniamo ai conti dello Stato - anche se non li approviamo - di consentire l'approvazione dopo una maratona notturna. La vostra risposta, ancora una volta arrogante e irresponsabile, è quella di dire: cari senatori, il PNRR, il piano da 270 miliardi (o quanti sono), voi non lo potete vedere e non lo potete discutere perché abbiamo già deciso tutto noi; anzi hanno deciso tutto loro: il Consiglio dei ministri o quella parte del Consiglio dei ministri che decide che cos'è il PNRR e il futuro del nostro Paese. E, come nei momenti più bassi della storia delle istituzioni, i senatori sono stati compensati con una pioggia di emendamenti puntuali per finanziare i provvedimenti da 7.000 euro, come neanche nel più sperduto consiglio comunale di campagna. *(Applausi)*. Questo è il Senato della Repubblica! Se a voi va bene, a noi non va più bene e non intendiamo tacere ancora. È una cosa che non è più tollerabile. Protestiamo con tutte le nostre forze rispetto al fatto che non ci è consentito di fare il nostro dovere di senatori. Signor Presidente, la nostra richiesta, ancora una volta, è quella di discutere di questi argomenti, che voi considerate decisivi e di cui vi riempite la bocca in ogni occasione nei convegni, in televisione nei *talk show*, dopo Natale

la nostra protesta sarà non partecipare a un dibattito a cui non possiamo dare il nostro apporto per il semplice fatto che voi ci impedite di portare il nostro contributo. Un contributo deve essere motivato, studiato, frutto di riflessioni, di un confronto anche all'interno del nostro Gruppo, ma tutto questo è impossibile voi lo avete deciso. L'unica opposizione responsabile presente in Parlamento ha il dovere di ricordarlo, per cui noi non parteciperemo a un dibattito finto di un Senato che ha rinunciato a svolgere il proprio ruolo e lo diremo in tutte le occasioni. Il nostro unico intervento sarà sulla questione di fiducia

so che è inutile - i colleghi di maggioranza a ripensarci e a fare un esame di coscienza: domandatevi se quello che ho detto è vero o è falso, se è frutto di partigianeria politica o di un'osservazione oggettiva della realtà politica di questo Paese. Ho concluso e ribadisco la nostra richiesta di calendarizzare l'esame del decreto-legge sul Piano nazionale di ripresa e resilienza dopo Natale.

Comprendiamo il rammarico e comunque anche il tema che ha posto il il Gruppo Fratelli d'Italia, perché - questo lo diciamo più volte al Governo - anche il fatto di aver affrontato PNRR e manovra di bilancio in contemporanea, pur dividendoli tra Camera e Senato, ha penalizzato fortemente il lavoro del Parlamento e ha messo in difficoltà fortemente il lavoro degli stessi uffici della Ragioneria e del Ministero dell'economia e delle che non sono stati messi nelle condizioni - così come ci è stato detto - per i tempi troppo stretti, addirittura di lavorare sugli emendamenti che i Gruppi politici avevano concordato. Ci siamo trovati per la prima volta

è una cosa che davvero non mette il nostro Paese in grandissima luce davanti a tante altre situazioni.

ci è stato chiesto di dare gli emendamenti prioritari in tempo utile, salvo poi arrivare all'ultimo minuto e dire che non c'era più il tempo di lavorarci. Quindi, il Governo avrebbe il compito di programmare in modo migliore i provvedimenti importanti che arrivano in Parlamento, per dare la possibilità al Parlamento stesso di fare il Parlamento: questo è l'elemento importante che noi sottolineiamo. Quindi, comprendiamo le rimostranze che il Gruppo Fratelli d'Italia ha messo in evidenza. È altrettanto vero che conosciamo - l'abbiamo detto tutti, Fratelli d'Italia compreso - l'importanza dei fondi che arriveranno dall'Europa; motivo per cui, scadendo il decreto sul PNRR il 5 gennaio, o comunque avendo una scadenza molto vicina, abbiamo la necessità di essere responsabili e andare verso l'approvazione del provvedimento. La Commissione oggi avrà tutto il tempo necessario per esaminarlo

il lavoro l'abbiamo fatto tutti e non veniamo qua a dare lezioni ad altri. Questo deve essere chiaro. Sul calendario - mi permetto e concludo - abbiamo accolto l'invito del Governo:

Facciamo però il possibile come Governo, nonostante sia programmata la giornata del 24, perché i tempi si stringano e il Parlamento possa arrivare alla votazione della legge di bilancio

Signor Presidente, anche noi in questi giorni complicati, in cui in Commissione bilancio si è deciso il testo di questa norma, abbiamo fatto, ovviamente nel nostro ruolo di maggioranza, quello che i colleghi di Fratelli d'Italia stanno facendo ora nel loro ruolo di opposizione. Abbiamo chiesto al Governo quello che sostanzialmente chiediamo dall'inizio di questa legislatura a tutti i Governi che si sono avvicendati in quest'Aula: chiediamo di metterci in condizione di fare la nostra parte, di fare il Parlamento e di non assistere in maniera passiva al passaggio di norme che cambiano l'aspetto del nostro Paese e la vita degli italiani. Ci abbiamo provato e il Governo che è qui sa che ciò che abbiamo discusso durante queste giornate non è stato banale. Abbiamo discusso del metodo,

maggioranza e opposizione. Concordo con il collega Romeo nel dire che l'opposizione è stata molto comprensiva e diligente nello svolgere la sua funzione di opposizione costruttiva; un'opposizione che comunque si è confrontata sui contenuti, ha presentato i suoi emendamenti e ha avuto soddisfazione per una parte di essi, come è giusto che sia. Anche l'opposizione rappresenta, infatti, una parte del nostro Paese. Quindi, per quanto ci riguarda, ciò che dice il collega Ciriani non è solo opportuno, ma è anche doveroso. Purtroppo, però, non so se le modifiche che sono state fatte all'interno di questo Emiciclo, sulla struttura, sul numero dei senatori,

Ciò che è stato fatto in questa legislatura, in questi anni, in queste ore, in questi giorni e sarà fatto nelle prossime ore,

legge. È un compito che tutti noi, come maggioranza e opposizione, ci dobbiamo assumere, perché tutti noi dobbiamo rispondere di quello che facciamo qui dentro ai nostri elettori. Ovviamente non mi permetterei mai di dare lezioni ad alcuno. È una constatazione che noi facciamo per la nostra parte. Ma credetemi - il Governo ci è testimone - per noi non è stato facile passare attraverso un processo di discussione ed elaborazione di una legge di bilancio che molto spesso ci ha fatto fare dei sacrifici metodologici e contenutistici. *(Applausi)*. Abbiamo però fatto la nostra parte, come è doveroso fare in un momento in cui, ancora una volta, non sono finite l'emergenza sanitaria e quella economica, non è finita, ma anzi si è implementata, l'emergenza sociale. Questa è la nostra posizione, Presidente, e questo il motivo per cui, al netto di ogni ipocrisia, noi di Forza Italia chiediamo, e ci abbiamo pensato, quanto sposterebbe trasferire la discussione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da domani a dopo Natale, posto che comunque il 31 dicembre dovrà essere approvato e posto che tutti noi siamo consapevoli del fatto che non possiamo modificarlo. Questo, però, ritiene e pertiene alla patologia di cui prima parlavo: non la presenza, ma la portanza dell'organo parlamentare. È un problema che prescinde dai numeri e che dovremo affrontare tutti insieme come classe dirigente del Paese. Tutto ciò premesso, per non farla troppo lunga, Presidente, condividendo le perplessità, ma assumendoci tutte le responsabilità, come Forza Italia ha sempre fatto dall'inizio della legislatura, noi chiediamo che venga confermato il calendario deciso in Conferenza dei Capigruppo, pur se a maggioranza. Speriamo che, in occasione della discussione

per evitare che ciò che è stato affrettato, ciò che ha rappresentato uno strappo, che noi abbiamo in qualche modo rabberciato, non diventi uno strappo ancora più profondo.

Signor Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, nel mio intervento parlerò di agricoltura e lo farò perché nella manovra di bilancio purtroppo se ne è parlato poco, molto poco rispetto a un settore non solo primario per definizione, ma fondamentale per la nostra economia, dove l'agricoltura e l'agroalimentare rappresentano un quarto del nostro PIL. Non se la prenda il ministro Patuanelli, cui vanno tutta la mia stima e simpatia personale, ma non si può sbandierare il fatto che in questo disegno di legge di bilancio le risorse per l'agricoltura siano raddoppiate rispetto alla precedente legge quando, in termini assoluti, su una manovra di quasi 30 miliardi di euro, non si arriva che a poche centinaia di milioni come risorse dirette per il settore. Parlo di risorse dirette: meno forse del 2 per cento. Signor Presidente, non è solo una questione di fredde cifre. Questi numeri dimostrano quanto poco centrale sia l'agricoltura nell'agenda politica di questo Governo, che di fatto dimostra di non credere, perché non investe e non dedica risorse, non dico importanti, ma almeno accettabili a un settore che, in questo periodo di crisi dovuta alla pandemia, ha dimostrato di non arrendersi mai e di garantire il cibo per tutti, compito non facile nell'attuale contesto.*(Applausi)*. Ma ci sono altri elementi che ci preoccupano, Presidente. Il primo è fondamentale e determinante per la tenuta del settore. Abbiamo l'impressione e sinceramente ce ne dispiace - che non ci siano una visione, un piano strategico per la nostra agricoltura, ma che si cerchi di mettere sempre una toppa alle troppe emergenze; tante tappe e nessuna visione. Una mancanza di visione - a nostro avviso - si registra anche nella mancanza, ad oggi, di un piano strategico nazionale, da presentare fra pochi giorni alla Commissione europea per l'attuazione della prossima Le Commissioni in Parlamento ad oggi non sanno cosa ci sia scritto in quel documento. Non sappiamo, perché il documento non è passato da queste sedi, quali siano le priorità, gli indirizzi, gli obiettivi, i mezzi. Insomma, non sappiamo, al di là dei contorni, quali siano le azioni cui si vuole spingere la nostra agricoltura. Chiudo la parentesi sulla PAC e non entro nella questione del PNRR, che già è stata ampiamente illustrata dal nostro capogruppo Ciriani. Ci dispiace per alcune polemiche di qualche amico, collega senatore, ma io credo che approvare questo Piano - come è stato detto invece che domani, la prossima settimana, è vero non avrebbe cambiato nulla nella sostanza, ma avrebbe permesso a tutti noi senatori di avere una prontezza rispetto a quanto vi è scritto. Si parla tanto di transizione ecologica. Sento che i colleghi se ne riempiono molto la bocca, signor Presidente. I *leader* europei lanciano *slogan* che sicuramente colpiscono l'immaginario collettivo: 3 miliardi di alberi da piantare da oggi al 2030. Siamo già in ritardo, perché ad oggi non se ne è piantato, di fatto, nemmeno uno. Ma, se proviamo a fare un conto veloce, significa piantare 300 milioni di alberi l'anno, un milione di alberi al giorno. Ma ci rendiamo conto? Vi rendete conto, colleghi senatori, di cosa stiamo parlando? Ma ammesso - e non concesso - che sia anche possibile, mi chiedo - e lo chiedo al Governo - se esiste un piano di piantumazione nel nostro Paese. Ma soprattutto, chi produce questi alberi e quanti se ne possono produrre? Non lo sappiamo, perché non c'è alcuna strategia.

Non solo: la legge sul florovivaismo, approvata alla Camera ed esaminata in Commissione agricoltura, è bloccata in Commissione bilancio dai primi giorni di agosto. siamo in piena transizione ecologica e la legge sul settore vivaistico è bloccata da mesi, dalla Ragioneria dello Stato, che ha espresso un parere negativo su un testo già approvato da un ramo del Parlamento, di fatto, di votare tutti quegli emendamenti che sicuramente avrebbero migliorato il testo. Insomma, abbiamo bisogno di piante e blocchiamo una legge per dare certezze a chi le produce. Rimaniamo sempre sul tema ambientale, Presidente: stiamo attraversando una vera e propria emergenza relativa alla fauna selvatica, che sta mettendo a serio rischio l'equilibrio faunistico e ambientale. È soprattutto un fenomeno che sta mettendo in ginocchio molti agricoltori e allevatori. Potrei parlare per ore, descrivendo la moltitudine di fauna selvatica che danneggia l'agricoltura, ma è chiaro che il più eclatante è il fenomeno del sovraffollamento dei cinghiali, che ormai arrivano a passeggiare tranquillamente nelle strade delle città.

Per fortuna, non si è ancora verificato un caso di attacco alle persone. I cinghiali sono un pericolo per l'ambiente, ma soprattutto un pericolo sanitario. Questi animali

Si stanziano risorse per la sterilizzazione, invece di predisporre risorse per un serio piano nazionale straordinario di abbattimenti, al fine di portare quegli animali a un numero sostenibile, per poi mettere in campo tutte le azioni necessarie per il contenimento, compresa la modifica della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ormai vecchia di quasi trent'anni e non più idonea ad affrontare le situazioni odierne. Non si mettono risorse per compensare gli agricoltori da questi danni.

A parte il caso della legge sul florovivaismo, mi si vuole spiegare perché, quando c'è un provvedimento che funziona (penso all'agricoltura 4.0), deve scendere in campo la contabilità per depotenziarlo solo perché drena risorse? crea sviluppo, economia e occupazione va mantenuto e - anzi - potenziato. Purtroppo, però, siamo in uno strano Paese: se qualcosa funziona, meglio abolirlo o modificarlo per renderlo meno appetibile.

Mancava un sostegno al comparto della birra, da supportare con adeguate risorse e una maggiore semplificazione normativa, soprattutto per agevolare il settore della birra artigianale. Per fortuna, con gli opportuni emendamenti abbiamo in parte risolto la questione. Abbiamo proposto una proroga dell'entrata in vigore del registro di carico e scarico dei cereali, per rendere più facile e comprensibile le relative procedure per aiutare la filiera in questo difficile momento. Peccato aver trovato un muro da parte del Governo.

previste risorse per compensare i danni da fauna selvatica, di cui ho già detto. Ne approfitto, però, per ricordare a quest'Assemblea e a lei, signor Presidente, che esiste una relazione finale su un atto assegnato,

è stata prevista per la gestione delle risorse idriche, che diventano fondamentali in questo sistema climatico sempre più imprevedibile.

Il sistema climatico può mettere in crisi molte produzioni e far perdere la qualifica di produttore agricolo a causa della perdita della prevalenza della produzione. Per fortuna, almeno in questo, il Governo ci ha voluto ascoltare. Allo stesso modo, ha ascoltato l'appello legato alla rinegoziazione del debito.

per tutelare i nostri pescatori e, automaticamente, i nostri mari dall'assalto selvaggio di flotte e pescherecci di altri Paesi che certamente poco rispettano le regole imposte ai nostri pescatori. Niente: ci dispiace

mediazione al ribasso e di cercare di accontentare tutti, il che non fa certo bene alla Nazione. Soprattutto, però ritengo - e lo ribadisco - che l'agricoltura ha bisogno di una visione che, da questa legge di bilancio, certamente non appare.

un po' di attenzione perché credo di dover dire delle cose abbastanza importanti. Mi dispiace che l'Assemblea non sia rappresentata al massimo, perché parlerò delle prerogative del Parlamento e del ruolo dei singoli parlamentari, approfittando della discussione del disegno di legge di bilancio, sul quale

del superbonus, della proroga delle cartelle esattoriali, del reddito di cittadinanza così come modificato, della magistratura onoraria credo che sia un passo importante per cercare di trainare definitivamente il Paese fuori dalle secche. Si poteva fare di più, si poteva fare di meglio; sicuramente il Parlamento avrebbe potuto incidere maggiormente, ma abbiamo fatto ancora una volta prevalere gli interessi del Paese a quelli territoriali e dei singoli partiti. In questa sede desidero, però, segnalare un antipatico episodio che si reitera da parte del Governo nei confronti del singolo parlamentare. Nel decreto-legge sostegni fu approvata una norma che modificò temporaneamente, quindi non a sistema, la legge sugli appalti, consentendo agli imprenditori morosi con il fisco non soltanto di partecipare alle gare (mentre la legge sugli appalti ne prevedeva e ne prevede la esclusione), ma addirittura la sospensione delle procedure esecutive. Da quel momento il sottoscritto ha cercato di introdurre in tutti i provvedimenti che si sono succeduti una norma priva di copertura finanziaria e che non era in contrasto con il sistema, una norma conseguenziale a quella modifica che era stata fatta nel decreto-legge sostegni. Quell'emendamento affermava che, se è vero che gli imprenditori morosi non soltanto vedevano sospese le procedure ma potevano partecipare alle gare di appalto, a maggior ragione l'avrebbero potuto fare coloro che invece durante le gare avevano addirittura estinto il loro debito. Questo emendamento nei vari provvedimenti ha trovato sempre un'opposizione, e non per motivazioni politiche - io l'avrei capito - ma per motivazioni tecniche da parte di funzionari, capi dell'ufficio legislativo, consulenti e non so chi altri dei Ministeri, che hanno accampato motivazioni inconsistenti, ingiustificate, irrazionali. E si è arrivati, signora Sottosegretaria, alla discussione del decreto-legge fiscale, in cui il Sottosegretario che rappresentava il Governo, in una infuocata discussione - non so quanti colleghi erano presenti nelle Commissioni riunite 6a e 11a - mentre rischiava di andare in minoranza su questo emendamento, propose l'approvazione di un ordine del giorno.

a questa ingiustizia e irragionevolezza - che riprendeva esattamente l'ordine del giorno sul quale il Governo aveva espresso parere favorevole. Si è trattato, quindi, non soltanto di un atteggiamento ostruzionistico, ma anche di una mancanza di lealtà nei confronti dei parlamentari. Su questo emendamento ancora una volta si sono inseriti i soliti noti, che hanno espresso un infondato parere. Io vi prego di valutarlo. Leggo Leggo delle dichiarazioni sibilline del presidente Draghi. Lui dice che pensa al presente e non al futuro e dice anche che il Governo andrà avanti senza di lui. Io chiedo formalmente al presidente Draghi, in virtù del mandato popolare che ho ricevuto e in virtù di quell'impegno che ho sottoscritto nel febbraio del 2021, sostenendo questo Governo, se è cambiato qualche cosa rispetto alle prospettive che si era dato. Chiedo, cioè, se ha intenzione di continuare a portare avanti il Paese verso l'uscita dal tunnel o se, invece, in presenza del

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

perché, praticamente, molti senatori hanno portato a casa dei micro emendamenti: qualcosa che non si era mai visto. visto. Veramente, voi, che siete il Governo dei migliori, siete per noi il Governo dei migliori a cambiare ciò che servirebbe agli italiani in favore del territorio con queste micro spese, che naturalmente possono portare consenso sul territorio. Noi credevamo di averle viste già tutte, invece ci mancava la legge mancia. mancia. È proprio una vagonata di micronorme. Non le leggerò, anche perché non so quanti di voi abbiano letto veramente, visti anche i tempi molto compressi,

Colleghi, il linguaggio è una convenzione. Le parole hanno un peso. Voi usate l'espressione manovra espansiva: intanto, vorrei fare una precisazione. Se si potesse parlare, al netto delle marchette, di manovra espansiva, questo Governo non avrebbe nessun merito. La manovra espansiva è determinata dal PNRR, quindi dalla montagna di soldi che arriveranno. Peraltro, come ha detto molto bene il nostro capogruppo, senatore

questioni per gli italiani, per la montagna di soldi che arriveranno, voi non date nessun tempo di leggere e di approfondire. Ma non mi dilungo su questo, perché il capogruppo Ciriani è stato

siate in grado di spenderli, e, dall'altra parte, della sospensione del Patto di stabilità. Pertanto, non arrogatevi davanti agli italiani dei meriti, che non sono vostri. Vorrei ora ragionare su due questioni: da una parte, il metodo e, dall'altra parte, il merito. Sul metodo, siete riusciti a fare peggio di qualsiasi Governo. Questa legge di bilancio arriva nettamente in ritardo al Senato, ma soprattutto è stata bloccata per più di un mese in Commissione bilancio. Voglio essere chiara perché non vorrei mai che gli italiani pensassero che la colpa del ritardo di questa approvazione sia dato all'opposizione. No, non

la legge di bilancio perché ognuno aveva una bandierina da portare a casa, al netto degli interessi degli italiani. Questo è il motivo del ritardo; questo è il motivo per il quale siamo ancora qua oggi ad aspettare. Certamente noi non avremmo votato la fiducia. Una Una volta c'era vergogna se veniva posta la questione di fiducia sul disegno di legge di bilancio, perché giustamente la si considerava una delle leggi più importanti

Avremmo avuto una grande occasione con questo disegno di legge di bilancio. Fratelli d'Italia, come opposizione patriottica e responsabile, ha fatto di tutto per poter migliorare

Grazie a Fratelli d'Italia, finalmente ci sarà l'aerazione meccanica controllata nelle scuole. Tutti i giorni si parla della tragedia del Covid-19. Presumiamo - queste almeno sono le notizie di stampa - che domani o dopodomani ci sarà un'altra stretta del Governo anche per coloro che come me, la maggioranza degli italiani, hanno fatto la terza dose di vaccino: probabilmente scopriremo tra ventiquattro ore che anche chi ore che anche chi ha fatto la terza dose di vaccino dovrà farsi il tampone, il contrario di quello che avevate detto poche settimane fa, cioè che i tamponi non erano utili. Sappiamo, non perché lo dice Fratelli d'Italia, ma perché lo dice tutta la comunità scientifica, che i maggiori *cluster* sono nelle scuole e sul trasporto pubblico. Allora, anziché continuare a dire no, che è molto più facile che lavorare e trovare delle soluzioni, voi continuate su quella strada. Grazie a Dio, una cosa vera per combattere il contagio l'avete messa nella vostra legge mancia perché Fratelli d'Italia ha insistito, perché abbiamo visto che il nostro governatore delle Marche ha avuto grandi risultati con l'aerazione meccanica controllata. Questo è per dire che non siamo qua a fare un bieco ostruzionismo perché vogliamo essere contro. No, noi vorremmo essere a favore dell'Italia e degli italiani; vorremmo essere a favore di tutte le leggi che vengono fatte e che migliorano la qualità della vita delle persone, delle aziende e dei lavoratori, ma per voi forse è un discorso troppo complicato. Lasciatemi dire che non bisognava certamente scomodare una persona autorevole e di chiara fama come il presidente Draghi per fare una legge di bilancio così modesta, una legge di bilancio che non ha visione, che fa perdere una grande occasione agli italiani per consolidare questa ripresa,

egoisticamente - non parlo di tutti gli italiani, ma di tutti i senatori e i deputati - certi di poter fare un'ottima campagna elettorale. Auguri a questo Governo e a questa maggioranza. Noi siamo diversi e ne siamo orgogliosi. *(Applausi)*. Grazie questa legge di bilancio è la seconda dall'inizio della pandemia e, se quella dello scorso anno aveva a che fare soprattutto con l'urgenza di tamponare la crisi, questa deve avere l'ambizione di introdurre riforme strategiche di cambiamento, che siano collegate al grande piano europeo Next generation EU, che abbiamo fortemente voluto, e alle priorità del nostro Piano nazionale di ripresa e di resilienza. La pandemia ci ha colpito in maniera così forte perché la nostra era ed è una società troppo fragile e troppo divisa da ingiustizie e diseguaglianze. Abbiamo bisogno di riforme, non fini a se stesse, ma che raccolgano le istanze sociali, che correggano le storture che la pandemia ha mostrato impietosamente. Storture che sono un fatto politico, a cui dobbiamo dare una risposta politica, cambiando le cose rispetto a come erano prima, costruendo un nuovo modello di sviluppo che metta al centro la persona e il lavoro proprio nel momento in cui la rivoluzione delle tecnologie, degli algoritmi, dell'intelligenza artificiale reclama l'esigenza di un ruolo più forte della politica per dare voce a chi è invisibile o a chi si percepisce come invisibile. infatti, lavori e ci sono vite intere che per le nostre leggi è come se non esistessero. Uno di questi è il lavoro creativo e culturale delle arti performative e dello spettacolo. La pandemia ha colpito più duramente su questo terreno perché questo mondo, così complesso e frammentato, non solo è stato chiuso

Eppure intorno a noi continua a essere un momento non solo difficile, ma per tantissimi drammatico con il rischio di perdere intere generazioni di artisti e di tecnici. Li cito insieme perché è un unico mondo, un'unica filiera. C'è una dispersione professionale che costa moltissimo al nostro Paese, perché cultura e spettacolo sono la rappresentazione dell'Italia nel mondo e sono allo stesso tempo un formidabile moltiplicatore di sviluppo, crescita economica e occupazionale, idee, futuro, legami e coesione sociale. Sono una delle forme vitali e indispensabili della nostra democrazia; è l'Italia, amata e riconosciuta nel mondo per le sue arti. Eppure tutto ciò ha un prezzo alto e spesso inaccettabile, perché poggia sul vuoto del mancato riconoscimento È per questo che chiediamo di introdurre finalmente in Italia uno statuto sociale dei lavori delle arti performative e creative che riconosca a tutti tutele in caso di malattia e di maternità, che riconosca assicurazioni, previdenza e la possibilità di crescere la possibilità per il lavoro creativo di diventare impresa culturale e creativa, con dei sostegni specifici. L'emergenza non finirà finché non avremo cambiato un sistema che oggi è ingiusto. L'emergenza c'era già prima della pandemia, ma si faceva finta di non vederla. Per far cessare l'emergenza non bastano misure tampone, misure *una tantum*, che pure sono importanti nell'immediato, ma che rischiano di essere un sostegno conservativo che alla fine avvantaggia chi è già più forte. Serve, invece, una riforma strutturale che innanzitutto riconosca tutte le professioni (in un mondo che sta cambiando continuamente per le innovazioni digitali e in cui si affermano nuovi lavori e nuove tipologie) per fare in modo che nessuno rimanga fuori da un sistema universale di tutele. E per farlo la prima urgenza è riconoscere finalmente il carattere discontinuo del lavoro creativo; discontinuo perché l'arte e la tecnica artistica, per compiersi, hanno bisogno di un tempo di studio, di ricerca, di azione, di preparazione, di aggiornamento professionale. Questo tempo preparatorio è un lavoro, va riconosciuto come lavoro e va remunerato. Oggi, in questa legge di bilancio un primo passo, un fondo di 70 milioni di euro; è un primo passo, anche se non ancora sufficiente, perché servono e serviranno molte più risorse. Però è un primo riconoscimento delle istanze di questi mesi e noi proveremo a indirizzarlo subito, già nella discussione della legge delega (che è in corso), verso la creazione di una vera e propria indennità di discontinuità che sia strutturale che sia perno per misure universali di *welfare* per tutte le tipologie contrattuali, sia autonome che subordinate, che sia perno per riconoscere finalmente a tutti i lavoratori del settore creativo la possibilità di avere un trattamento pensionistico. Oggi per un lavoratore dello spettacolo è difficilissimo raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione, a causa di un effetto distorsivo di norme capestro, per cui accade che il fondo dei lavoratori dello spettacolo presso l'INPS abbia un avanzo patrimoniale di 5 miliardi e 400 milioni. utilizziamo! Perché sono risorse frutto dei contributi dei lavoratori dello spettacolo e delle arti performative; queste risorse vanno redistribuite ai lavoratori dello spettacolo in termini di misure di *welfare* universali. Noi pensiamo che intorno al riconoscimento del lavoro, che è la prima riforma e che deve essere il centro di questa nuova progettualità, altri tasselli poi debbano marciare insieme. Per questo deve affiancarsi la legge che abbiamo proposto a sostegno delle imprese, dei luoghi e degli spazi della cultura e dello spettacolo. Pensiamo ai *live club*, ai piccoli teatri di prossimità e di quartiere, ai centri culturali; c'è anche qui il riconoscimento di un sistema imprenditoriale e produttivo, ma insieme il riconoscimento di una rete di comunità e di presidio sociale che cambia vite e che tiene in piedi quartieri e città. Questa, Presidente, è una sfida tutta politica; non è una vertenza di categoria, ma è una sfida decisiva per l'intero sistema Paese,

perché non potrà esserci ripresa economica senza una visione politica, non potrà esserci protezione senza emancipazione. Questo lo dobbiamo in particolare alle nuove generazioni e a chi di più a chi di più sta pagando questa crisi. Per fare in modo che mai più nessuno si senta e sia invisibile. *(Applausi)*.

vorrei innanzitutto ringraziare tutti coloro che in questi ultimi giorni e in queste ultime notti hanno lavorato senza sosta per portare a termine l'esame degli emendamenti al disegno di legge gli uffici dei Ministeri, che hanno lavorato ai pareri e alle riformulazioni, anche se non sempre ci sono piaciute, anche se qualche emendamento, come quello a prima firma del collega senatore Floris sui lavoratori di Air Italy, ha avuto parere contrario (questa non è stata una bella notizia), anche se sulla rottamazione-*ter* e sulle rate scadute e non pagate il 14 dicembre non è stato fatto nulla, nonostante gli ordini del giorno presentati al decreto fiscale e nonostante tanti contribuenti non siano riusciti ad adempiere nei termini. Ringrazio i colleghi della Commissione bilancio, il presidente Pesco, i relatori, i Capigruppo e tutti i membri del Governo che hanno partecipato alle sedute. Sì, è vero, sono stati approvati diversi emendamenti localistici, settoriali, talvolta definiti in altro modo, spesso denigratorio, ma non sono tutti emendamenti da denigrare, né da sminuire nella loro importanza. Spesso, dietro un emendamento territoriale o settoriale c'è il lavoro di tanti uomini e di tante donne, quindi la vita di tante famiglie. Tutti sappiamo che è importante salvare anche una sola vita. Penso all'emendamento sui lavoratori portuali, alla proroga dell'indennità di mancato avviamento per i lavoratori dei porti di Taranto e di Gioia Tauro. Penso soprattutto al via libera alla costituzione dell'agenzia per il lavoro portuale per i lavoratori del porto canale di Cagliari: un grande risultato per cui ringrazio i colleghi sardi che hanno firmato con me l'emendamento o che hanno presentato emendamenti analoghi. Ringrazio la vice ministra Alessandra Todde per il lavoro svolto a monte. Sicuramente le famiglie di questi lavoratori trascorreranno un Natale meno triste e con un po' di speranza in più. Non ci sono solo piccoli emendamenti settoriali, ma anche grandi temi: l'avvio della riforma fiscale, con la riscrittura delle aliquote Irpef e l'abolizione dell'IRAP per le persone fisiche titolari di partita IVA. Quest'ultima è una conquista enorme voluta dal Parlamento, in particolare dalle Commissioni finanze di Camera e Senato, voluta dal MoVimento 5 Stelle. La riscrittura delle aliquote Irpef ha determinato una riduzione dell'Irpef soprattutto per quei contribuenti che vengono definiti ceto medio, ma che ceto medio non sono. I maggiori benefici in termini percentuali sono rivolti assolutamente alle classi di reddito più basse; i maggiori benefici in termini assoluti a chi prende uno stipendio attorno ai 2.000 euro mensili: lavoratori dipendenti, quella categoria che costituisce il 38 per cento dei contribuenti, ma che paga oltre il 50 per cento dell'Irpef complessiva e che non ha mai ricevuto benefici degni di nota in termini di riduzione dell'Irpef. Chi guadagna 2.000 euro al mese è sicuramente più fortunato di chi ne guadagna 1.800, ma non è ricco, soprattutto se ha famiglia, figli e mutuo: in questi casi, ahimè, si avvicina molto alla povertà. L'intervento che è entrato nel disegno di legge di bilancio va visto come una prosecuzione del taglio del cuneo fiscale che abbiamo introdotto nel 2020 e che prevede un *bonus*, un trattamento integrativo di 1.200 euro annuali, 100 euro mensili in favore dei lavoratori dipendenti con un reddito fino a 28.000 e e che dopo i 28.000 decresce fino a 40.000. Quindi, in realtà abbiamo pensato a tutti. Poi, Presidente, c'è il superbonus. Non voglio ripetere quello che hanno già detto i colleghi; questo è il più grande risultato che abbiamo ottenuto: salvare il superbonus per le case singole, eliminare la soglia ISEE di 25.000 euro Una proposta - quella scritta nel testo iniziale del Governo - che sarebbe stata discriminatoria e inaccettabile perché sarebbe andata a discapito soprattutto di chi vive nei piccoli Comuni dove la casa singola non è una villetta, come ci è stato raccontato in questi ultimi mesi, ma semplicemente una casa, è la casa. la casa. Vorrei dire un'altra cosa: il superbonus non è solo una misura straordinaria, non è solo una bandierina; non è solo una vera e propria politica economica, sociale ed ambientale che, nonostante tutti i tentativi di frenarla e di depotenziarla, nonostante le difficoltà iniziali, ci ha già permesso di raggiungere risultati enormi in termini di risparmio energetico, come è stato recentemente certificato dal CRESME. Il superbonus è qualcosa di più. Una delle caratteristiche dell'Italia è sicuramente il fatto che oltre l'80 per cento dei cittadini possiede una casa di proprietà, vive nella sua casa di proprietà. Questo è un elemento che sicuramente ci ha permesso di superare con minore apprensione le gravi crisi che abbiamo attraversato negli ultimi anni; sicuramente ci ha consentito sempre di essere più indipendenti e meno ricattabili rispetto a queste grandi crisi, Una misura come il superbonus ci renderebbe meno ricattabili anche rispetto alla crisi che ci attende in termini di approvvigionamento energetico e di costo dell'energia. Tuttavia, ci viene trasmesso, in maniera più o meno velata, il messaggio secondo cui avere le case di proprietà sarebbe un elemento in qualche modo negativo, da correggere e in ogni caso da punire. da punire. Ebbene, vorrei dire ai colleghi, al Governo e soprattutto all'Europa che avere una casa di proprietà e tenere alla propria casa non è una colpa o un peccato, è un gesto d'amore non solo per noi stessi, ma anche per la nostra famiglia, per le nostre compagne, per i nostri compagni, per i nostri figli; è il più grande gesto d'amore perché esprime tutta la premura e tutto l'interesse che abbiamo per il loro futuro. Quando rendiamo la casa ancora più bella, anche più calda, più protetta, più efficiente, non lo facciamo pensando soltanto all'aspetto economico, pur importante, ma pensando che in quella casa ci vivono e ci vivranno i nostri figli e vogliamo che ci vivano bene.

Signor Presidente, vorrei iniziare con un ringraziamento a tutti i colleghi della Commissione bilancio, al Presidente, ai relatori e ai tecnici che hanno supportato i i colleghi nel complesso lavoro di elaborazione degli emendamenti e della loro votazione. Siamo di fronte ad una legge di bilancio

senza tagli alla spesa pubblica. Si tratta di una legge di bilancio nella quale il Partito Democratico si riconosce pienamente, ricca di misure che rispecchiano ed interpretano l'impegno di un'importante forza politica riformista e progressista di centrosinistra. Le misure proposte, sono state sostenute nelle fasi di elaborazione, approvazione ed emendazione a livello di Commissione.

Sulla scuola abbiamo risorse per un dimensionamento scolastico triennale, per la stabilizzazione dei docenti e per il personale ATA, oltre che per le scuole paritarie: misure che ci stanno molto a cuore e sulle quali ci siamo impegnati. Ci sono misure importanti che riguardano i giovani, con norme e risorse per il contrasto al bullismo, per combattere il disagio psicologico, ma soprattutto che riguardano il potenziamento dell'apprendistato, con un freno agli *stage* non retribuiti e quindi un percorso di stabilizzazione del lavoro e di valorizzazione delle competenze dei giovani.

nostro emendamento, c'è un potenziamento del Fondo per la non autosufficienza, e poi ancora misure che riguardano le donne con finanziamenti per i centri antiviolenza e misure specifiche per gli uomini maltrattanti.

dei sindaci al fine di ridare dignità e riconoscere l'importante ruolo che i primi cittadini svolgono all'interno delle nostre comunità. Ci sarebbe piaciuto che venisse approvata anche la norma che riguardava

un riconoscimento di ruolo anche dal punto di vista economico. Cito inoltre i contributi pensionistici per i giovanissimi sindaci, che quando iniziano a ricoprire tale carica spesso devono abbandonare il lavoro, soprattutto se non hanno un'occupazione stabile, e si vedono privati della contribuzione pensionistica. Ci sarà modo anche in Commissione di proseguire questo lavoro che ci sta a cuore. C'è una copertura per quanto riguarda la TOSAP per i Comuni: ancora tre mesi gratuiti per l'occupazione di suolo pubblico per ambulanti

saputo ricomprendere molte delle misure che stavano a cuore al Partito Democratico. Una nota però sul metodo: ieri il relatore Errani ha opportunamente affermato che qualcosa è diventato patologico e pone un problema significativo di funzionamento della politica rispetto a come si è giunti all'approvazione in Commissione del disegno di legge di bilancio e alle difficoltà che ci sono state nel coordinamento di tutti i lavori. Credo che il tema sia davvero la politica; il sistema è inceppato e questa modalità di di funzionamento, che ormai è diventato un monocameralismo alternato perfetto, è di fatto una modifica della Costituzione materiale del Paese. La politica deve avere la capacità di affrontare la questione, non possiamo andare avanti in questo modo. Vi è la necessità di interrogarsi e di porre all'ordine del giorno una reale riforma costituzionale, che modifichi sostanzialmente le nostre modalità operative. C'è la necessità C'è la necessità di rivedere anche le regole di funzionamento parlamentare e i nostri Regolamenti, perché la presentazione di 6.200 emendamenti, quando il disegno di bilancio arriva già con un mese di ritardo, crea un ulteriore inceppamento del nostro meccanismo e non aiuta certo ad accelerare. una questione di forma: con tutto quello che ho detto prima e le difficoltà di metodo che abbiamo avuto, la presenza del ministro Franco oggi forse sarebbe stata opportuna. Ho grande stima della sottosegretaria Cecilia Guerra, ma la presenza del Ministro dell'economia quest'oggi sarebbe stata un segnale decisamente migliore rispetto al lavoro che abbiamo condotto tutti insieme.

desidero anticipare un ragionamento, che farò poi anche in dichiarazione di voto, perché questo disegno di legge di bilancio è particolarmente importante per tre aspetti: il è il fronte delle transizioni, il secondo è il fronte delle riforme, il terzo è il fronte dell'equità. Sul fronte delle transizioni, questa legge di bilancio si pone esattamente al fianco del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alimentando con risorse e norme quelle transazioni digitali, ecologiche, ma soprattutto sociali in cui ci siamo impegnati e che vede il nostro orizzonte di azione molto ravvicinato, al 2026. È un disegno di legge di bilancio importante per la sua portata: 23 miliardi su 30 sono alimentati dal *deficit* non è quasi mai successo. Sapevamo che con le clausole di salvaguardia il Parlamento e il Governo avevano 5 o 6 miliardi da utilizzare per rinnovare il Paese; invece, questo disegno di legge di bilancio utilizza uno spazio enorme, 23 miliardi, per rinnovare il Paese. Lo fa con coraggio, come sul fronte della riforma fiscale: è un primo passo nella riforma fiscale. In questo disegno di legge di bilancio si affronta il tema dell'Irpef, risolvendo quel problema storico, annoso, noto a tutti i tecnici del settore, che riguardava l'applicazione e i salti di scaglione, rendendo più equa la tassazione, alleggerendola moltissimo sui redditi medi e bassi. Lo fa anche facendo un primo passo per risolvere quell'imposta particolarmente iniqua che è sempre stata l'IRAP, abolendola per tutte le persone fisiche che non si vedranno più gravate da un'imposta ingiusta, ma soprattutto si vedranno totalmente escluse da ogni tipo di Il secondo fronte affrontato questi 23 miliardi è quello dello sviluppo economico e della transizione energetica. Ci sono misure molto importanti, sicuramente la più importante è quella dei bonus edilizi. Li abbiamo prorogati, abbiamo reso le norme fruibili, abbiamo fatto in modo in Parlamento che ci fosse un legittimo affidamento da parte di coloro che avevano iniziato i lavori e che avevano programmato di svolgerli, senza che venissero penalizzati rispetto a chi aveva iniziato e pensato di iniziare i lavori prima. È un passo avanti, un passo importante. Questa legge fa molto anche sul fronte dell'equità; introdurre infatti l'ammortizzatore unico universale, come aveva proposto già nella scorsa legislatura la senatrice Parente, in un interessante e approfondito disegno di legge,

sul fronte dei giovani. Abbiamo però molto insistito perché ancora una volta fosse prorogato e alimentato di risorse l'apprendistato, uno strumento importante per mettere i nostri più giovani e talentuosi ragazzi italiani nelle condizioni di iniziare a lavorare e di entrare nel mondo del lavoro. Molto ancora sui più fragili: ci sono risorse importanti sulla disabilità e un pacchetto di riforme alimentate anche da risorse sul tema dell'autismo. Risponde a delle criticità note, come quella della crisi sanitaria che ancora una volta ci vede tutti i giorni

che alimenta la bolla dei prezzi, a sua volta alimentata anche e purtroppo dai bonus edilizi. Lo fa però adeguando i prezzari rendendo le opere più efficaci e non utilizzabili per alimentare ulteriormente la bolla dei prezzi. in questo breve intervento è ciò che è stato inserito nel disegno di legge di bilancio su un fronte rispetto al quale si fanno molti convegni, ma nella pratica si mettono poche risorse e si scrivono poche norme. Mi riferisco alla parità di genere nel nostro Paese. Questa legge di bilancio fa dei passi fondamentali sul fronte dell'*empowerment* femminile, rifinanziando tutte le politiche in questo senso, mettendo però la nuova norma della certificazione aziendale sulla parità di genere nelle condizioni di essere efficace, facendo cioè in modo che tutte le aziende d'Italia siano pronte a certificarsi in termini di parità e portino le donne a poter lavorare molto oltre quello scarso 50 per cento che ci vede ultimi nella classifica europea con oltre 20 punti di *gap* rispetto non solo gli uomini, ma anche a tutte le donne europee. Fa molto sul fronte della violenza, una drammatica piaga italiana che vede oltre 6 milioni di donne coinvolte nel corso della loro vita. Viene rifinanziato il reddito di libertà per rendere le donne che hanno subito violenza capaci di riprendere in mano la propria vita e di percorrerla con forza, in libertà e con la possibilità di ricrearsi una vita libera dalle violenze. Viene fatta una riforma molto importante sul fronte della violenza

per il suo essere una legge non ideologica, ma molto equilibrata.

tante lacune, tante - mi si permetta il concetto puro della parola - deficienze, mancanze del nostro Paese. Il nostro Paese manca oggi di un sistema infrastrutturale, che è fragile, sia sotto il profilo stradale che sotto il profilo ferroviario; ha un sistema sanitario sicuramente considerato - e lo è in alcune parti - un'eccellenza, rispetto soprattutto ad altri Paesi, ma che ha mostrato grandi fragilità con il problema del Covid-19; un sistema di riforme in continua rincorsa, che dovrebbe essere in assoluto declinato in modo meno frettoloso; un sistema fiscale che viaggia con normative a tampone; un sistema di economia circolare ancora embrionale; un sistema economico e produttivo

anziché essere, nella sua natura, un provvedimento che rinforza un sistema base che dovrebbe essere già ben strutturato, diventa semplicemente

"cerotto", perché, con i suoi emendamenti, piccoli, grandi, diversificati, di contenuto più forte per alcuni e più leggero per

prossime ore, un altro provvedimento importante, che dovrebbe essere il provvedimento della ripresa oltre che della resilienza, il PNRR, ci troviamo a legittimare una serie di contenuti che sono fondamentali

questa situazione, perché effettivamente si potrebbe anche lavorare insieme, come abbiamo fatto (perché abbiamo lavorato in sinergia), ma con uno spirito sinceramente più costruttivo e soprattutto più incisivo. Cosa dire, ancora, di questo bilancio, oltre ai numeri che sono evidenti, alle alle diverse sfaccettature che gli emendamenti portano e a quello che ho già detto? Possiamo dire che ci saremmo aspettati la possibilità di interagire, come Gruppo parlamentare, in modo più forte.

fiducia nel vostro Parlamento. Noi, che siamo diversi e proveniamo da territori ed estrazioni politiche e culturali diverse, siamo comunque capaci di lavorare.

Non abbiamo bisogno di un atto schema da riempire con semplici criteri, di piccoli emendamenti che poi vanno compressi o di piccoli gruzzoli da distribuire come piccole mancette.

posizioni personali che, all'interno delle forze politiche, possono esserci, anche comprensibilmente. Tante forze politiche che oggi sono al Governo, per gran parte della legislatura sono state all'opposizione e, quindi, hanno condiviso con noi la stessa visione

far convergere tutti e che si arrivi un po' in ritardo, però tengo anche a stigmatizzare quella che non dev'essere e non deve diventare una prassi, che peraltro è peggiorativa di anno in anno,

Non credo che voi dobbiate concedere a noi degli emendamenti, anche perché, contrariamente ad altre proposte di modifica che prevedono magari assunzioni di due dipendenti in un Comune o ad emendamenti da 7.000 euro, come alcuni di quelli che compaiono in questa manovra, noi non ci siamo dedicati ad emendamenti *ad personam* o a gruppo; ci siamo dedicati a emendamenti che avevano un forte interesse generale, per i quali c'era grandissima condivisione dell'Assemblea. Non erano emendamenti di Fratelli d'Italia, per Fratelli d'Italia; erano emendamenti che ritenevamo necessari e condivisibili per riuscire ad incidere su questa manovra e a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, secondo il mandato che abbiamo ricevuto, come voi e come tutti. pertanto che anche il rispetto delle forze di opposizione si manifesti attraverso i fatti, ma anche attraverso le parole. mi dispiace sentir dire che qualcuno ci ha concesso di vedere approvati alcuni emendamenti, anche perché magari sono gli stessi che hanno chiesto di appoggiare i loro quando invece la maggioranza ne voleva appoggiare altri.

Se infatti fino alla legislatura scorsa la fiducia era un esproprio del Parlamento e qualcosa per cui attaccare costantemente il Governo Governo e doveva essere solo una misura straordinaria, cui si faceva ricorso solo nel momento in cui non era possibile fare altrimenti, voi avete istituzionalizzato il ricorso alla fiducia. Avete istituzionalizzato, dopo averlo osteggiato,

Non esiste più per la vostra prassi antidemocratica, senza il mandato di nessuno. Anzi, per una cospicua parte di voi, cioè per il partito di maggioranza relativa di questo Parlamento, è stata proprio la lotta al voto di fiducia, al voto di fiducia, contro l'antidemocrazia del Parlamento precedente, che vi ha consentito di rappresentare un terzo dei cittadini. Quindi, se c'è qualcuno che deve fare un esame per prendere un patentino, quelli siete voi: si chiama esame di coscienza e non avete bisogno che ve lo facciamo noi, lo potete fare tranquillamente da soli. È vero. Ho il massimo rispetto per quegli 11 milioni di cittadini italiani che vi hanno dato fiducia. Hanno anche la mia massima solidarietà, solidarietà, totale ed estesa. Non sono più 11 milioni, perché, oggettivamente, i sondaggi ci dicono che sono molti di meno, ma ce l'hanno, perché hanno creduto di votare qualcosa e si sono trovati in realtà Noi, invece, con la massima responsabilità e con la massima lucidità di chi ha usato magari toni forti, ma non si è mai posto contro le istituzioni (nessuna!), neanche quando le occupate voi, voi, abbiamo mantenuto e continuiamo a mantenere sempre, come unico faro, l'interesse nazionale, anche quando l'unico faro e l'unico interesse che avete voi è continuare a rimanere qui a occupare questi banchi. Signor Presidente, ho chiesto la parola per denunciare, ancora una volta, l'anomalia democratica che si consuma in questo Parlamento. Il bicameralismo è finito e al suo posto abbiamo un monocameralismo notturno. Tutti noi abbiamo assistito in questi giorni alla prassi insana di decidere le sorti del Paese durante la notte, come i fuggiaschi, con continue convocazioni della Commissione bilancio per ben 15 volte, dopo il termine fissato al 29 novembre per la presentazione degli emendamenti: praticamente un *record*, nella stagione del monocameralismo di fatto. Cos'è questa, se non la volontà di esautorare la funzione dei parlamentari e di questa nobile istituzione? Dare corso a decisioni già prese dal Governo e dal Governo e ad accordi a porte chiuse. Chi si è rifiutato di obbedire a questa prassi è stato, ovviamente, tagliato fuori. Molti nostri colleghi si sono lamentati per la perdita di dignità. Sono passati solo alcuni emendamenti. La cosa più grave, tuttavia, non è questa, ma lo spettacolo che abbiamo dato al Paese. Avevo presentato, assieme ad altri colleghi, un emendamento per consolidare l'*iter* dei livelli essenziali delle prestazioni. LEP non possono limitarsi alla sola assistenza sociale, annunciata in pompa magna ieri, come se bastasse solo quella per colmare il divario dei servizi. I livelli essenziali delle prestazioni costituiscono invece il perno per trovare finalmente una soluzione alla disuguaglianza territoriale che attanaglia da decenni il nostro Paese, che anche l'Europa stigmatizza. È vero che nella manovra si fa riferimento per la prima volta ai LEP e potrebbe essere un passo avanti, se non fosse che, come denunciato da pochi colleghi, ciò viene fatto in maniera annacquata, senza un cronoprogramma né un ancoraggio certo al fondo di perequazione e, soprattutto, senza che nessuno conosca il testo del mitologico disegno di legge sull'autonomia differenziata. Il mio emendamento sui LEP mirava in sostanza a rafforzare la funzione del Parlamento (la sua "portanza", è stato detto in Aula), chiedendo il parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni delle due Camere e della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, stabilendo che il Governo, prima di istruire qualunque atto per rispondere a richieste delle Regioni, si presenti prima alle Camere per chiedere un atto di indirizzo, al fine di limitare l'arbitrio di Governo e Regioni. Proponevo inoltre di cancellare il riferimento ai costi *standard* e di specificare che la spesa *pro capite* per ciascun servizio - lo sottolineo - dev'essere uguale su tutto il territorio nazionale, fatta salva la necessità di predisporre azioni perequative a favore dei cittadini di aree attualmente svantaggiate come quelle del Mezzogiorno. Cosa è stato di quell'emendamento? Non è dato saperlo, perché si è deciso tutto nottetempo. Questa mossa fa il paio con quella concertata di decidere su altri tavoli, ignoti al Parlamento, il testo mitologico del disegno di legge sull'autonomia differenziata. Che cosa significa? Significa che alcune Regioni non soltanto otterranno più competenze, ma manterranno un maggiore gettito fiscale nei loro territori, violando così i principi di solidarietà e unità della Repubblica sanciti dalla nostra Costituzione. Il Parlamento però ha deciso chi gestisce queste risorse? Le gestirà il Ministero? Le gestiranno le Regioni o altri soggetti istituzionali? Diversamente, si rischia infatti di creare "repubblichette" che minano alla radice l'unità nazionale. Tra l'altro, la pandemia ha dimostrato con chiara evidenza che la regionalizzazione di risorse e competenze - vedi la sanità - non è garanzia di efficienza, ma l'esatto contrario. Dunque, non è per niente vero che l'autonomia, come dice qualche governatore del Nord, fa bene a tutti; fa bene solo agli interessi di qualcuno. Lo schema è chiaro ed è inquietante per noi, ma gli italiani non lo sanno, perché non viene detto loro, né dalla politica, né dalla stampa, e non si discute nel Parlamento, né dentro, né fuori dalle istituzioni. È vero che è stato accolto l'ordine del giorno a mia firma sull'autonomia differenziata e sui LEP

ma, se un ordine del giorno è una stretta di mano tra gentiluomini, adesso sta al Governo tenere fede alla parola data, accogliendo l'ordine del giorno. Rimane il fatto che con

Signor Presidente, onorevoli senatori e rappresentanti del Governo, la legge di bilancio rappresenta sempre uno degli appuntamenti più importanti, anzi il più importante in assoluto, al quale Parlamento e Governo sono chiamati ogni anno. In questo 2021 però la manovra è tanto più importante perché, insieme al PNRR, deve rappresentare un punto di svolta e di ripartenza rispetto alla drammatica esperienza del Covid. La pandemia infatti, oltre alle ovvie ed evidenti ripercussioni di carattere sanitario ed economico alle quali questa manovra vuole dare una risposta, ha avuto ripercussioni tragiche anche dal punto di vista sociale, soprattutto per quanto riguarda il suo effetto sui minori. I più piccoli devono essere sempre destinatari di un'attenzione particolare e tanto più è giusto che lo siano adesso, dopo aver vissuto lunghi mesi particolarmente duri che, tra *lockdown*, periodo di chiusura delle scuole e altre limitazioni, ne hanno minato la socialità e in molti casi hanno provocato veri e propri disagi, a cui è indispensabile dare risposta immediata. L'impossibilità di incontrarsi con gli amichetti o i cuginetti, di andare al parco giochi o anche di fare una semplice passeggiata al parco ha avuto effetti devastanti sui bambini. Da Presidente della Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza mi sono attivata perché venissero approvate misure nell'interesse dei più piccoli.

È infatti proprio la sua pervasività a rendere il cyberbullismo tanto più grave e pericoloso del bullismo, perché, tra *smartphone*, *social network* e *app* di messaggistica, questa vera e propria piaga non abbandona i ragazzi praticamente mai. Non c'è dubbio che la pandemia, soprattutto nei mesi in cui le scuole erano chiuse e i ragazzi comunicavano solo con i *social*, abbia acuito questa problematica, che ha conseguenze drammatiche, rendendoli insicuri, impauriti, spaesati e perlopiù incapaci di reagire. La prevenzione passa necessariamente dalla conoscenza e dalla capacità di individuare un fenomeno subdolo come quello del cyberbullismo. È proprio per questo motivo che ho proposto l'istituzione di un fondo *ad hoc*, così che genitori, insegnanti e associazioni del settore possano essere adeguatamente formati per riconoscere e quindi porre un freno a questo tipo di abuso e soprattutto per aiutare chi ne è vittima. Si tratta di una battaglia che, con l'intera Commissione, conduco da anni e che, con l'istituzione di questo fondo, compie finalmente un fondamentale passo in avanti. Parimenti, la centralità di ragazzi e bambini trova nuova linfa attraverso un'altra proposta che vedrà la luce con la legge di bilancio: il finanziamento con 2 milioni di euro dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, un'istituzione fondamentale che, grazie a questi stanziamenti, potrà finalmente svolgere il suo ruolo in maniera pienamente operativa, con un proprio organico e una struttura capace di affrontare l'impegnativo lavoro che quotidianamente è chiamata a svolgere. Ritengo poi semplicemente fondamentali i soldi destinati dalla manovra alla figura dello psicologo nelle scuole. Come dicevo all'inizio, il Covid ha infatti avuto ripercussioni gravissime sulla socialità e sul benessere psicofisico dei ragazzi, tanto più con la didattica a distanza che per mesi ha inchiodato gli studenti davanti a un *monitor* o a uno *smartphone*. I dati fanno rabbrividire: il suicidio è diventato la seconda causa di morte tra i ragazzi dai quindici anni in su, mentre gli episodi di autolesionismo anche tra i bambini sono aumentati del 45 Sono numeri spaventosi, che ci fanno comprendere quanto sia indispensabile fornire un sussidio psicologico adeguato ai nostri ragazzi, anche presso una delle due principali agenzie educative, ovvero la scuola. Da mesi si discute della necessità di convincere gli indecisi a vaccinarsi, ma mai finora ci siamo posti il problema del timore che potrebbero avere anche i più piccoli nel momento in cui i loro genitori decidessero di vaccinarli adesso. Ebbene, sono certa che nei prossimi mesi il ruolo dello psicologo a scuola sarà utilissimo anche rispetto all'esigenza di tranquillizzare i bimbi *under* 12 in attesa di vaccinarsi o subito dopo aver ricevuto il vaccino. Oltre alle misure di cui ho appena parlato, trovo poi assolutamente positiva l'introduzione del *bonus* con cui si intende far fronte ai disturbi mentali, perché sappiamo che le ricadute di questa pandemia sono molteplici e spesso molto gravi, tanto da necessitare di un sostegno adeguato, che non tutti possono permettersi. Da qui la decisione di sottoscrivere un emendamento a prima firma collega Gallone, presentato anche da altri Gruppi, proprio a salvaguardia della salute mentale che per molti è stata messa a dura prova in questa pandemia con le varie restrizioni. Non ci sono che due modi per superare l'incubo che stiamo vivendo da due anni: possiamo possiamo soffermarci a guardare le macerie che questa pandemia sta lasciando dietro di sé oppure possiamo reagire, sfruttando al meglio i mezzi che abbiamo a disposizione. Ogni misura è perfettibile e si può sempre fare di più e meglio, lo sappiamo, ma di certo non posso che esprimere enorme soddisfazione per l'attenzione che è stata dimostrata in questa manovra all'universo dei minori, destinatari di misure e di finanziamenti importanti, necessari ormai da molti anni; quindi, È iscritta a parlare la senatrice Lezzi. Ne ha facoltà.

Per quanto riguarda il taglio dell'Irpef, è stato importante un subemendamento voluto dalla Lega per la clausola di neutralità

per far sì che il caro bollette diminuisca e si trovi una soluzione, perché questo incide notevolmente sull'economia reale di tutti i giorni.

utilizzato solo in emergenza, perché l'obiettivo del Governo dev'essere quello di dare l'opportunità di trovare lavoro. Ben vengano quindi tutti i paletti che sono stati inseriti

Altro tema toccato è quota 100. La Lega ha battagliato perché le persone, soprattutto i lavoratori fragili e usuranti, possano continuare ad andare presto in pensione. Abbiamo ottenuto quota 102, anche se saremmo stati più contenti di poter continuare su quota 100:

sì, per sostenere la famiglia, ma dev'essere anche riconosciuto quello che è stato fatto nel corso della vita, quindi con una giusta ed equa pensione ai nostri cittadini.

TOSAP e COSAP: è evidente che nel periodo pandemico bisogna cercare di dare la possibilità agli esercenti e ai conduttori di pubblici esercizi di lavorare anche all'esterno. È importante anche il fondo turismo, con 150 milioni, 150 milioni, per poter dare sostegno a coloro che sono stati più colpiti quest'anno. Sicuramente sono stati fatti i vaccini, chiediamo i tamponi per le persone che vengono dall'estero, ma mi raccomando: non possiamo più permetterci di chiudere, abbiamo una stagione invernale davanti e dobbiamo fare in modo che i nostri operatori possano continuare a lavorare. La montagna ha già pagato un caro prezzo l'anno scorso, abbiamo la necessità di lavorare e di continuare a far vedere i nostri bellissimi territori anche ai Paesi esteri. Vorrei aggiungere un ulteriore tema per il territorio, visto che ho parlato di turismo: è stato approvato un emendamento che crea un fondo

del tempo sospeso, perché, se ci volgiamo alle nostre spalle e al passato recente, troviamo una condizione complicata e difficile, ma, anche se guardiamo avanti, il tempo rimane sospeso, perché il futuro, pur migliore rispetto

all'inizio della riforma fiscale, dall'intervento per calmierare l'aumento delle bollette all'accelerazione che vi è stata - ed è un merito di questo Governo e del suo Capo - nel nel contenimento della pandemia. Vorrei ricordare il Presidente del Consiglio e il generale Figliuolo per le attività che hanno messo a disposizione di questa straordinaria Italia. Eppure, c'è bisogno oggi di un'accelerazione che riguardi la vaccinazione dei più piccoli. Non sono più ammessi ritardi e temo che presto debba essere presa in considerazione anche l'obbligatorietà del vaccino, per evitare che l'emergenza parziale nella quale viviamo possa diventare strutturale. Si indicano due pilastri che vengono rafforzati e il disegno di legge di bilancio, da questo punto di vista, fa il paio con il *recovery

Quello che invece manca e dovrebbe essere valorizzato ancora di più è ogni forma di intervento contro la povertà, che è destinata ad allargarsi e fa il paio con l'emergenza, che non è ancora scomparsa. Dobbiamo avere a cuore le sorti dei più deboli e di chi è rimasto indietro, per molte ragioni, e, non da ultimo, per una decisiva: se le istituzioni perdono la capacità perequativa perequativa e di redistribuire, quel che resta della democrazia parlamentare va in crisi e prevalgono forme pericolose di sovranismo nazionalista. Lo sappiamo già: la sfiducia genera paura e dalla paura germina l'antipolitica. Non possiamo permettercelo, in una fase così delicata.

e l'aprile 2021, per fronteggiare a vario titolo e in vario modo l'emergenza pandemica, il Governo ha impegnato una cifra che è pari a circa 179 miliardi di euro in tredici Lo dico per mettere nella giusta considerazione e nella giusta cornice la cifra del superamento di una fase delicata, quella pandemica, dell'emergenza piena del 2020 e in parte del 2021, con le tante speranze che affidiamo al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta di due cifre non equivalenti, ma con molti puntini di sospensione. Temo, signora Presidente e Governo, che ci sia necessità

che seguì la Seconda guerra mondiale, la ricostruzione postbellica. Allora lo si fece confidando in una Italia cristiana e legata alla terra, che lavorava dall'alba al tramonto e che oggi non c'è più. È un'Italia che va riscoperta perlomeno però per i valori di base, che sono, da una parte, quelli della solidarietà umanitaria e, dall'altra, la creazione di un fronte repubblicano che si ponga l'obiettivo di creare rete fra le Istituzioni, a cominciare dal Parlamento. Invece il Parlamento, signora Presidente, è assente in maniera preoccupante. Vorrei dire peggio che assente, quando stiamo discutendo di una legge di bilancio quale chi ha una qualche esperienza parlamentare - e io sono fra questi - non può citare alcun tipo di precedente. Nessuno. Ricordo soltanto un numero:

40 leggi su 80 hanno avuto il voto di fiducia, che avremo di nuovo domani, addirittura bino, uno probabilmente nella tarda mattinata o nel primo pomeriggio, l'altro probabilmente nella notte o nella mattinata di venerdì.

evocato e invocato il ritorno alla democrazia parlamentare e alla logica della piena rappresentanza non perché il Parlamento in sé debba essere centrale, ma perché il Parlamento in sé è il luogo della rappresentanza politica e istituzionale più alta e, come tale, richiede rispetto. Il Parlamento è invece in un angolo e non è soltanto un problema di emergenza pandemica.

un'esagerazione di individualismo e la somma di questi due fattori, alla fine, è la paura e l'assenza della speranza, cioè la solitudine e l'isolamento di chi soffre di più e dei più deboli. Si risponde anche nel modo che ho provato ad indicare. Immagino che l'elezione del Capo dello Stato debba essere un punto di partenza e non il punto centrale di un'equazione soltanto parlamentare. Se posso fare un esempio, citerei quello di Einaudi, che rappresentò l'inizio della fine di un ventennio, a Costituzione appena approvata, e l'inizio di una Italia che si avviava a diventare felicemente democratica. Siccome in quest'Aula, Presidente, si è parlato addirittura della tutela del sughero nazionale e siccome il Parlamento europeo si sta avviando a discutere del proprio futuro e del futuro dell'Unione europea, quanto mai utile sarebbe una sessione parlamentare da destinare a discutere apertamente e coralmente del futuro dell'Italia. Continuo a pensare

Signor Presidente, colleghe e colleghi, intervengo oggi per sottolineare il segnale dato dal Gruppo Partito Democratico, dal Senato e dal Governo ai nostri connazionali all'estero.

Già la Commissione di cui mi onoro di far parte, nella stesura del parere, aveva dato il segnale di un convinto sostegno alle nostre comunità all'estero. Con l'approvazione della legge di bilancio, stiamo dando contezza a un lavoro svolto in maniera certosina e soprattutto di enorme valore, Due milioni di euro vengono aggiunti agli investimenti dell'Italia per le nostre comunità all'estero. Per la promozione della lingua e della cultura italiana sono stati stanziati 600.000 euro aggiuntivi rispetto al finanziamento a regime, destinati in particolare al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura nelle scuole locali. Per il personale a contratto presso le rappresentanze diplomatiche e consolari sono stati stanziati 800.000 euro a decorrere dal 2022, quindi in maniera permanente, per adeguare le retribuzioni. Infine, per il sostegno alla rete dei consoli onorari, sono stati stanziati 600.000 euro, un ulteriore segnale alla rete di servizi per le nostre comunità, che ha subito forti pressioni in questi anni a causa dell'emergenza sanitaria. I consoli onorari, infatti, facilitano l'accesso ad importanti servizi ai nostri connazionali che vivono lontani dalle sedi diplomatico-consolari. Immaginate il caso degli italiani che vivono a Darwin, in Australia, ad oltre 3.000 chilometri dal consolato di Brisbane. Entriamo nel merito di questi tre importanti interventi. È stato ribadito il forte interesse dell'Italia per i nostri connazionali fuori confine e per una maggiore proiezione del sistema Italia nel mondo, grazie al sostegno dei programmi per la diffusione di lingua e cultura. Il nostro Paese si arricchisce e si espande nel mondo, anche - e, direi, soprattutto - con la diffusione della sua lingua Un ulteriore sostegno va a favore di quanti ogni giorno sono impegnati a garantire i servizi della rete consolare all'estero, gli impiegati a contratto, che rappresentano un'importante parte del motore dell'amministrazione oltre confine. Tanti fattori hanno guidato la nostra azione politica per l'approvazione di risorse per un adeguamento dei loro salari. Fra questi ricordo la conclamata carenza di personale e l'oggettiva vacanza di organici, l'aumento del costo della vita nei Paesi della rete diplomatico-consolare, le tensioni sui mercati dei cambi e un netto peggioramento delle condizioni di vita, legato al progressivo deterioramento del quadro internazionale, che si riverbera in un aumento dei fattori di rischio e disagio. Risultati come questi vanno a beneficio della rete consolare, ma soprattutto delle nostre comunità e dei servizi che ricevono ogni giorno. Sempre nell'ottica della garanzia di maggiori servizi ai nostri concittadini all'estero, sono stati stanziati ulteriori fondi per la rete dei consoli onorari, che operano soprattutto nei Paesi in cui si trovano le più alte concentrazioni delle collettività italiane o in quelli interessati da intensi flussi turistici, dove spesso sono richiesti interventi a tutela dei connazionali in difficoltà. La presenza *in loco* di un console onorario può essere, in molti casi, risolutiva di diverse problematiche. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha da tempo avviato un progetto volto a dotare i consoli onorari delle attrezzature per la rilevazione dei dati biometrici per il rilascio di passaporti. Tale progetto, oltre ad essere visto favorevolmente dalla collettività, ha consentito un notevole risparmio di tempi e costi, ma si è tradotto in un ulteriore onere, spesso pesante, per i consoli onorari. Voglio ricordare che i consoli onorari ricevono solo un contributo per il rimborso spese, che in molti casi ha solamente un valore simbolico, a fronte delle significative spese che sono tenuti a sostenere. Il contributo previsto in questa manovra di bilancio è un risultato importante e un segnale verso coloro che ogni giorno sono impegnati, a vari livelli, a sostegno dei servizi ai nostri concittadini nel mondo. Come accennato all'inizio, tanti sarebbero stati i temi da trattare, tutti importanti, ma - purtroppo - non è stato possibile affrontarli. Voglio qui ricordarne due, secondo me lasciati in sospeso e che hanno bisogno di una particolare attenzione: il primo riguarda la rete delle camere di commercio italiane all'estero e il secondo il valore del turismo di ritorno. Spero che nei prossimi provvedimenti, ma soprattutto nell'attuazione dei progetti del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, questi due temi possano entrare nell'agenda e nei programmi di investimento. Le camere di commercio italiane nel mondo sono connesse a rete, in un sistema di promozione radicato sui territori che costituisce un punto di riferimento per le comunità di affari locali e un supporto di servizio alle piccole e medie imprese italiane. rappresentano un *network* istituzionale in grado di offrire informazioni di prima mano e servizi di accompagnamento nei diversi mercati e hanno svolto e continuano a svolgere un grande lavoro per l'*export* italiano e per attrarre investimenti in Italia. Il loro ruolo diventa ancora più importante oggi, per contribuire alla ripresa *post* pandemia. Hanno bisogno di rilanciare le proprie attività con rinnovato entusiasmo ed energia, ma la pandemia ha purtroppo prodotto danni significativi. In molti casi riescono a sopravvivere solo grazie al lavoro volontario degli associati e la speranza è che le cose possano cambiare nel futuro. Sarebbe non solo opportuno, ma necessario un impegno affinché vengano stanziate più risorse da investire nelle camere di commercio italiane nel mondo, nell'ambito dei progetti di internazionalizzazione,

Oltre il 15 per cento del turismo internazionale in Italia è costituito da persone di origine o discendenza italiana e costituisce il cosiddetto turismo di ritorno. Oltre a visitare le grandi città italiane, spesso si recano nei borghi dove sono nati loro o i propri genitori o nonni. È un segmento del turismo che dobbiamo valorizzare. Sarebbe auspicabile un impegno a maggiori investimenti, in particolare costruendo infrastrutture ricettive nei borghi e promuovendo iniziative a favore delle comunità italiane nel mondo che facciano conoscere le bellezze ambientali e storiche, la ricchezza delle tradizioni, la bontà della gastronomia e lo stile di vita salutare dei piccoli centri italiani. Tutto il Partito Democratico è impegnato su questi temi, in quanto si tratta di investimenti per il bene dell'Italia. Insieme ai colleghi eletti nel Partito Democratico alla Camera e al coordinamento del Dipartimento per gli italiani del mondo del PD, siamo sempre stati impegnati e continueremo a lavorare per il riconoscimento e la valorizzazione delle comunità degli italiani nel mondo.

per l'instancabile e convinto impegno. Gli investimenti dell'Italia di cui abbiamo parlato oggi sono il risultato di un lavoro di squadra che ha portato i suoi frutti e che dà un segnale positivo alle nostre comunità; è un ulteriore passo volto a valorizzare le nostre comunità nel mondo. Infine, signor Presidente, mi permetta di augurare a lei e a tutte le senatrici e tutti i senatori e alle loro famiglie buon Natale e felice anno nuovo.

il presidente Draghi è venuto in quest'Aula a chiedere la fiducia per il nuovo Governo, con la promessa che avrebbe fatto una grande rivoluzione fiscale. Sarebbe stata la riforma delle riforme, perché avrebbe dovuto concorrere finalmente alla crescita di questo Paese sulla spinta del PNRR. Da lì è partito il balletto di tutti i partiti, che in Commissione hanno presentato di tutto e di più, illudendo gli italiani che finalmente ci sarebbe stata una vera grande rivoluzione fiscale. Ci siamo trovati poi in Parlamento con una manciata di miliardi, non molto differente da quelli che ci sono sempre stati negli ultimi anni, anche in questa stessa legislatura.

significava essere davvero coraggiosi, e prevedere anche un'imposta negativa per chi ha meno. Voi invece siete andati al ceto medio, per il quale ho grandissimo rispetto, ma quando le risorse sono poche si pensa agli ultimi, agli ultimi, che adesso si ritrovano anche a barcamenarsi con l'aumento delle bollette. È curioso l'intervento della collega della Lega, che chiede di più in merito alle bollette. Eppure

se per i truffatori del reddito di cittadinanza non si arriva a 200 milioni, gli aumenti delle bollette possono arrivare fino a 14 miliardi. su questo meno di un terzo e state qui a compiacervi e a compiacere il *Premier,* che poi vi lascia le briciole su cui scannarvi in piena notte per i rifacimenti del parcheggio della chiesa vicina alla casa del senatore di una stradina comunale, in modo da poter ostentare un potere che non avete, perché siete ridotti a marionette *(Applausi).* Però è furbo e spietato Draghi: vi ha incartato per la prossima legislatura, perché forse nessuno di voi ha avuto il coraggio di leggere come poi si andrà a intervenire nella riduzione del debito. Quando sventolate la bandierina per la quale si potranno avere più mesi per pagare le cartelle esattoriali, vorrei vedere anche una levata di scudi, perché il sottosegretario di Stato alla Presidenza

ancora lascia a terra gli operai, stabilendo un bel percorso e prevedendo una sanzione che è addirittura conveniente per le multinazionali che potranno non far niente in quei tre mesi. Per darvi qualcosa vi stanno trattando da miserabili, questa è la verità, ma chi paga chi paga sono i poveri operai e le loro famiglie che si ritroveranno a piedi, ma con le vostre belle parole, le vostre belle banderuole. il Parlamento è diventato sostanzialmente inutile, ma subisce una sorta di umiliazione collettiva della rappresentanza. Oggi ho sentito il presidente Draghi dire che c'è stata la discussione. Fa una pessima figura il presidente Draghi. Lui, tra i più capaci, non è riuscito a presentare il disegno di legge di bilancio nemmeno nei tempi: è arrivato con un mese di ritardo. Poi vi ha lasciato qui in una sorta di limbo, perché non diciamo che il disegno di legge di bilancio è stato discusso. Non si è discusso assolutamente nulla: le sedute della 5a Commissione sono state convocate e sconvocate di continuo e qualche capo bastione di partito è andato in processione al MEF giusto per qualche mancetta, perché di questo si parla. Tutto il resto è stato tristemente deciso dal MEF. qualche parola sul lavoro, su quanto poco si stia facendo per il lavoro e quanto sia stato anche mortificato il reddito di cittadinanza. cittadinanza. Voi avete previsto una commissione e poi non l'avete ascoltata; una commissione che aveva messo l'accento sui *navigator*, i quali avevano trovato un deserto, dovuto sicuramente alla gestione trentennale dei centri per l'impiego, utilizzati come serbatoi di manovalanza,

nel frattempo avete allargato le maglie dei Ministeri, dove state assumendo e nominando di tutto e di più: da esperti esterni a funzionari. Avete allargato le maglie di tutto. Brunetta assume chi vuole, con il suo albo, mentre i *navigator* avevano fatto anche una prova selettiva, neanche molto semplice. Questi li state mandando via, così Brunetta fa le sue assunzioni. State abbandonando a loro stessi di percettori del reddito di cittadinanza, che avrebbe bisogno del pubblico, l'unico in grado di accompagnare costoro verso un vero inserimento nel mondo del lavoro,

a lavorare. Non avete voluto neanche guardarli gli emendamenti, dicendo: li abbiamo prorogati per quattro mesi. Se vogliono, è così, altrimenti se ne andassero a quel Paese. Questo è il succo del discorso. Ed è veramente mortificante che un Governo di unità nazionale, un Governo che dovrebbe agire davvero per il bene del Paese non abbia preso a cuore determinate situazioni.

Non c'è niente che trasformerà, che rivoluzionerà la vita della povera gente. Ricordo che la Lega

Bene, è il momento di tirarle fuori, perché le bollette stanno lì sul comodino e gli italiani avranno serie difficoltà. Brunetta, anche lui, aveva 50-60 miliardi pronti nel cassetto per fare la *flat tax*: tiratele fuori queste coperture, perché la gente lì fuori

Non credo che lei abbia capito e, quindi, necessita che io le spieghi. Io non l'ho interrotta nel corso di tutto il suo intervento, nonostante

ai partiti che, in questo momento, anziché pensare alle urgenze del Paese, hanno pensato a tutt'altro. Ora io vi faccio i miei migliori auguri. Quasi tutti voi potrete andare a spendervi i 100.000 euro, i 10.000 euro o i 15.000 euro sul territorio, per dire finalmente: avete visto? Sono un senatore potente! Ho portato i soldi, ho fatto il parcheggio della chiesa sotto casa. Bravi! Intanto, però, gli italiani avranno altro urgenze e voi li state di nuovo illudendo, senza risolvere assolutamente nulla, pensando sempre ed esclusivamente ai fatti vostri. Grazie Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, entrerò subito in argomento. Quale Italia - è stato chiesto - pensiamo per i prossimi decenni?

la politica devono discutere di questo. Il tema energetico e ambientale, pur vero e grave - siamo già in ritardo di anni e di decenni che si tramuta in transizione ecologica, dovrà essere graduale e compatibile con la situazione reale e dovrà essere studiato a fondo perché non è detto, ad esempio, che l'elettrico sia la soluzione. Saremo in futuro una Nazione manifatturiera, dove il fisco e la burocrazia consentono di produrre ricchezza o saremo soltanto la Nazione e vado per riassunto - del mandolino? Difenderemo le nostre produzioni nazionali a tutti i costi, anche rispetto all'Europa, quando ci attacca sul vino, sulle case o su altre cose? L'Istituto Bruno Leoni, illustre centro di pensiero di Torino, ha detto che siamo di fronte alla stagnazione produttiva pluridecennale dell'Italia. Siamo di fronte al problema dell'inflazione che, fino a certi limiti, è benefica, ma oltre va controllata, altrimenti è pericolosa per gli interessi e per i risparmi. Siamo di fronte alla conseguenze della pandemia che, oltre che dal punto di vista sanitario, ha causato quello che sappiamo sui prezzi e sull'energia. Il problema dell'energia deriva dal no alle centrali nucleari. Abbiamo deciso la riforma fiscale, che è un primo passo, ma che è fatta purtroppo per pochi miliardi, è stato detto, ma è fatta a debito e a debito non si risolve nulla, né per le famiglie, né per le aziende, né per lo Stato. I vincoli di bilancio sono saltati. Il rapporto tra *deficit* e PIL quest'anno è al 9,8, per cento, mentre è previsto per il 2022 in legge di bilancio al 5,6 il debito totale è a 2.700 miliardi (un anno fa parlavamo di 2.350-2.400 miliardi) e ci sono altri miliardi, compresi quelli del PNRR, che andranno aggiunti a questo importo mastodontico.

originario - vedremo poi nel maxiemendamento - sulla rivalutazione dei beni, che riguarda soltanto i marchi e l'avviamento; non è prevista la rivalutazione dei beni immobili e delle partecipazioni, ma, come si è sempre fatto,

sui crediti bancari fino al 30 di giugno nel settore dell'autotrasporto, che piange la concorrenza straniera o perlomeno di chi ha la sede in Romania. Pensiamo di risolvere tutto con lo *smart working* che fino al 3 o 5 per cento - e dico delle percentuali a naso - può essere utile e praticabile, ma oltre crea problemi al sistema di procedura delle ditte e, soprattutto, della

detto, ci avversa su tante cose e bisogna veramente battere i pugni. L'accordo con la Francia - è un mio grido di dolore in quest'Aula - è pericoloso, perché la settimana dopo l'accordo Macron è andato negli Emirati Arabi Uniti e ha fatto una commessa da circa 20 miliardi di elicotteri, sottraendola ad aziende nazionali. Una manovra a parte - una

bella intuizione, in qualche modo corretta rispetto alle previsioni iniziali dell'articolo 9, ma è partita su presupposti sbagliati.

sottolineato: in primo luogo la rimodulazione degli scaglioni e, in secondo luogo, la riduzione delle aliquote, proprio per cercare di aiutare il ceto medio,

quindi comunque i redditi bassi usufruiscono già di alcune agevolazioni. Dai 12.000 euro a salire, la rimodulazione delle aliquote, con l'intervento sulle detrazioni e l'assorbimento del *bonus* Renzi, fa in modo che tutti gli italiani avranno una riduzione delle tasse. Chi più e chi meno, a livello progressivo, perché questo è scritto nella nostra Costituzione, tutti avranno questa riduzione. Si tratta di un risultato chiaro ed evidente. L'altro risultato a cui teniamo particolarmente, perché è una battaglia storica della Lega, è aver ottenuto finalmente l'abolizione dell'IRAP per un milione tra ditte individuali, professionisti

di ditte individuali e professionisti ai due milioni che hanno beneficiato della mini-*flat tax*, introdotta quando la Lega era al Governo all'inizio della legislatura, arriviamo a 3 milioni di partite IVA, che erano state dimenticate per anni dallo Stato italiano. Grazie all'intervento della Lega oggi finalmente beneficiano di una riduzione delle tasse. Non saranno risultati epocali, ma - perdonatemi se ci rifacciamo sempre al pragmatismo - sono risultati concreti e tangibili che nessuno può negare. Non è tutto, però, perché la riduzione delle tasse è un pacchetto importante e fondamentale in questa manovra, ma ci sono stati anche altri interventi che reputiamo decisivi: 100 milioni di euro stanziati per il turismo, viste tutte le difficoltà di questo momento a causa del Covid, 50 milioni per il settore dell'*automotive* per cercare di aiutare le nostre imprese e i nostri produttori. Sono loro che devono essere aiutati; non serve solo una politica legata agli incentivi sulle auto, ma una politica rivolta alle piccole aziende. Noi siamo pieni di terzisti; c'è il mondo dei concessionari che è in notevole difficoltà e per loro abbiamo ottenuto un fondo importante.

che hanno subito le chiusure durante il periodo Covid e che sono stati in grandissima difficoltà. Questo è un risultato certo e condiviso da tutte le forze politiche. È un risultato che abbiamo ottenuto e di cui dobbiamo andare fieri. Potrei citare anche altre tematiche importanti come l'incremento di 27 milioni di euro del fondo per l'autismo. Questo è quanto ci aveva chiesto espressamente il nostro ministro Stefani

preoccupato di aumentare l'organico. È una battaglia fatta dal sottosegretario Molteni e da Salvini in primo luogo. *(Applausi)*. Se oggi abbiamo delle assunzioni di Forze dell'ordine insieme a una tutela legale è solo ed esclusivamente merito della battaglia e dell'impegno della Lega.

e riguarda i nostri allevatori. Sono risultati fondamentali, ma di certo non basta. C'è il tema delle bollette, che qualcuno ha evocato. Bisogna sterilizzare questo aumento delle bollette. Intanto il Governo ci ha messo 3,8 miliardi, che non è poco. Serve di più; siamo noi i primi a richiamare un tavolo che metta in campo ulteriori risorse, perché ci sono molte aziende che rischiano di chiudere e di mettere in pericolo la produzione.

va fatta con gradualità e intelligenza. Altrimenti saremo in testa a un treno, sulla locomotiva di un treno che va diretto a sbattere contro un muro, perché avrà costi altissimi in termini di posti di lavoro e in termini sociali per tutta la popolazione. Quindi tutela dell'ambiente sì, ma "gretinismo" no.

alla pandemia, ma al contempo sta continuando ad affermarsi una forte domanda di beni pubblici e di azioni pubbliche che riguardano tematiche quali l'ambiente, lo sviluppo sostenibile, la protezione sociale e il lavoro. Questi beni pubblici e queste azioni pubbliche non potranno che essere sostenute da massicci investimenti pubblici, come sta emergendo anche in Europa dopo il Next generation EU, i cui effetti daranno enorme beneficio all'Italia grazie all'iniziativa e agli sforzi del Governo Conte II, che l'ha ottenuto un anno fa. Ed è ancora grazie a quel Governo, all'intuizione e alla perseveranza del MoVimento 5 Stelle che oggi possiamo sottolineare l'avvenuta estensione e il potenziamento di una vera e propria rivoluzione qual è il superbonus 110 per cento per l'edilizia. di una misura innovativa basata sul meccanismo dello sconto in fattura e sulla cedibilità dei crediti d'imposta, introdotta proprio dal Governo Conte II nel maggio 2020, in piena pandemia. Voglio ricordare questo dato anche per sottolineare che quel Governo, con il costante *input* del MoVimento 5 Stelle, non solo ha saputo stendere una rete di protezione intorno al tessuto economico e sociale del Paese nel corso della pandemia, ma ha anche avuto la forza e la lungimiranza di puntare subito sul rilancio del Paese, mettendo in campo misure innovative che in pochi mesi hanno spiegato i loro benefici effetti. Dall'ANCE al CRESME, passando per l'ENEA, Unioncamere, le associazioni imprenditoriali, gli ordini professionali (e potrei continuare, perché l'elenco è davvero lunghissimo): nell'ultimo anno non c'è praticamente osservatore economico che non abbia certificato i grandi effetti del superbonus sulla crescita del PIL italiano ed europeo, sulla generazione di nuovi posti di lavoro, sull'apertura di cantieri e sul conseguimento di obiettivi di risparmio energetico e di tutela dell'ambiente. Ebbene, grazie al MoVimento 5 Stelle oggi riusciamo a estendere e a potenziare il superbonus. A partire dal testo originario della legge di bilancio abbiamo esteso il superbonus al 2023 sui condomini e sulle case popolari; le modifiche parlamentari che abbiamo richiesto a gran voce e ottenuto lo estenderanno per tutto il 2022 a beneficio delle case unifamiliari. Abbiamo così cancellato la precedente e sbagliata previsione di un tetto ISEE, ISEE, che avrebbe discriminato i cittadini e sarebbe stata del tutto incoerente rispetto agli obiettivi del superbonus, che sono quelli dell'efficientamento energetico e della messa in sicurezza antisismica. Così come abbiamo abolito il limite, precedentemente previsto, riferito all'abitazione principale (quindi lo si potrà fare anche per le seconde case), nonché il limite della presentazione di una CILA, addirittura retroattiva. Tutto questo l'abbiamo cancellato semplicemente perché era sbagliato. Un'altra modifica importantissima riguarda la proroga fino al 2025 del superbonus 110 per cento per gli interventi antisismici nelle aree che sono state colpite da eventi sismici a partire dal 2009 in poi (quindi i terremoti che hanno interessato le nostre Regioni italiane dal 2009 in poi). Inoltre, proroghiamo ed estendiamo la misura del superbonus agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, agli impianti fotovoltaici e alle colonnine elettriche di ricarica, comprendendo anche gli edifici di proprietà di ONLUS e di RSA. Questa misura, che contraddistingue così tanto questa legge di bilancio, dimostra quanto il MoVimento 5 Stelle sia fortemente schierato a difesa di uno dei beni più preziosi per gli italiani: la casa. Proprio attraverso questa misura, il superbonus, andiamo a proteggerla,

lo abbiamo sostenuto fin da subito noi del MoVimento 5 Stelle, attirandoci in qualche caso il sarcasmo dei soliti soloni della politica e dell'economia - che, per la verità, non ne azzeccano mai una - però, questo succede a tutti gli innovatori, quali noi crediamo di essere. Ora, dopo i risultati che sono stati certificati, di cui vi ho parlato prima, lo sostengono praticamente tutti, compresi il vice presidente della Commissione europea Frans Timmermans e la commissaria all'energia Simpson, che hanno enfatizzato gli effetti di questa nostra misura davanti al Parlamento europeo. L'intuizione del MoVimento 5 Stelle non si fermerà qui; il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito, vera ragione del successo del superbonus e dell'esplosione dell'utilizzo degli altri bonus edilizi, rappresenta una innovazione che si presta a essere estesa anche ad altri crediti di imposta, come quelli legati al nostro piano Transizione 4.0 che riguarda il settore produttivo, anch'esso confermato in legge di bilancio e reso triennale

La manovra è importante anche per un'altra operazione di rilievo, ovvero la diminuzione dell'Irpef, che dà un doveroso segnale a quel ceto medio che ha sempre puntualmente pagato la maggior parte delle imposte, senza finora avere mai una boccata di ossigeno. Allo stesso tempo riusciamo a dare un segnale importante anche alle fasce più basse, soprattutto nel combinato disposto della riforma dell'Irpef e la decontribuzione decontribuzione fino a 35.000 euro di reddito, l'assegno unico per i figli e il taglio al cuneo fiscale sui redditi bassi (quest'ultimo operato l'anno scorso dal Governo Conte 2). In questo disegno rientra anche lo storico azzeramento dell'IRAP per più di 800.000 partite IVA, che rappresentano oltre il 40 per cento dell'intera platea: operazione - questa - che era attesa e invocata da anni, ed è importantissima perché prelude al definitivo assorbimento dell'IRAP in un'imposta unica sulle società, che è uno degli obiettivi della delega fiscale all'esame del Parlamento. Mi avvio davvero alla conclusione, Presidente. Abbiamo ottenuto un miliardo in più per il reddito di cittadinanza, misura che durante la pandemia ha aiutato milioni di italiani, quelli più fragili e indifesi, i bambini, i disabili, gli anziani, che senza l'aiuto del reddito di cittadinanza sarebbero rimasti sprovvisti di protezione e avrebbero pagato un prezzo altissimo alla crisi. E pensare che diversi esponenti politici, anche in quest'Assemblea, hanno provato strumentalmente a evocarne l'abolizione o un taglio delle risorse ad esso dedicate, citando dati falsi,

sottolineo - dei percettori del reddito, quelli abili al lavoro, hanno firmato un contratto di lavoro; quindi, altro che fannulloni, altro che metadone di Stato o le volgarità che sono state dette.

Signor Presidente, farò una breve replica agli interventi che sono stati copiosi e ricchi di spunti per un disegno di legge di bilancio che ha accolto sicuramente molte istanze delle colleghe senatrici e dei colleghi senatori.

dai colleghi senatori e senatrici perché siamo riusciti veramente a destinare ottime risorse, ad esempio, per l'autismo, la qual cosa ci ha veramente dato soddisfazione, come spero darà molta soddisfazione alle persone che ne hanno più bisogno.

disegno di legge di bilancio: ad esempio, vi sono 150 milioni a disposizione di un fondo per la sostenibilità ambientale, che permetterà anche alle nostre industrie di riconvertirsi e pensare a un futuro migliore attraverso una nuova strategia legata a nuovi cicli di produzione e a nuovi sistemi di

ma bisogna riconoscere - e bene ha fatto il collega Quarto a ricordarlo - che per quanto riguarda la sostenibilità e la biodiversità c'è ancora tantissimo da fare. Soprattutto c'è da fare molto sul dissesto idrogeologico. A tale riguardo va apprezzato lo sforzo del MoVimento 5 Stelle volto a destinare risorse, minime ma importanti, per portare avanti la realizzazione della Carta geologica d'Italia, che è sicuramente uno dei fattori base per riuscire a fare di più, per migliorare l'assetto idrogeologico italiano ed evitare le catastrofi che copiosamente accadono anno dopo anno. Il collega Vitali ci ha ricordato una questione molto importante e che purtroppo in

per riuscire a ridurre le tasse ai cittadini. Sicuramente si potrà fare ancora molto di più migliorando il rapporto tra fisco e cittadini, attraverso l'informatica, la digitalizzazione, un rapporto più diretto e veloce con il fisco. Ad esempio, già riuscire a spendere in modo immediato e rapido le risorse destinate ai crediti di imposta potrebbe rappresentare un vantaggio per i cittadini: un portafoglio fiscale nel quale riuscire ad ad accantonare e spendere in modo veloce e rapido le risorse destinate ai contributi fiscali. Speriamo che questo possa diventare presto realtà; siamo molto fiduciosi. La collega Ronzulli ci ha ricordato l'importanza del supporto psicologico nelle scuole. C'è da fare sicuramente molto; un segnale concreto lo abbiamo dato

Il collega Perosino ci ha ricordato i problemi con il debito pubblico: bisogna fare sicuramente molto di più, lo sappiamo benissimo, ma lo si fa attraverso quelle misure, piccole o grandi che siano,

ma alla fine chi deve intervenire sono sempre le Forze dell'ordine. È un segnale molto importante il fatto che verranno assunte

una cosa vergognosa, ma vergognose sono anche le condizioni di lavoro degli agenti di Polizia penitenziaria, pochi

Questo ha mortificato oggettivamente il lavoro parlamentare e ha fatto bene la senatrice Faggi a ricordare che invece il Parlamento, che è fatto anche di tante competenze, intelligenze e conoscenze approfondite delle realtà territoriali, è una ricchezza per il Governo e non solo un passaggio dovuto.

del PNRR alla Camera, ci siamo trovati a lavorare in grandissima fretta; una fretta che ha colpito evidentemente anche i membri del Governo che hanno dovuto seguire i provvedimenti,

di fare degli errori. Ci sono infatti delle questioni sulle quali bisogna trovare il tempo di riflettere, e non un tempo infinito, ma il tempo di poter fare degli approfondimenti proprio per vedere la direzione nella quale si vuole andare insieme.

in tutte le sue sfaccettature è una delle attività più importanti del nostro Paese, che dà lavoro veramente a tantissime persone, nei vari ruoli.

che bisogna cercare di rendere più visibile possibile, più efficiente possibile e più accessibile possibile tutto il mondo del turismo. cioè migliorare davvero il Paese, ma soprattutto bisogna poi saperlo comunicare, perché il potenziale è così alto che possiamo diventare davvero il Paese di riferimento di tutto il mondo. Tutti devono avere desiderio di programmare una vacanza nel nostro Paese per la bellezza naturale, per la ricchezza del patrimonio artistico delle nostre città,

del senso critico delle persone, è un momento di divertimento. È un settore dove esiste tanta precarietà proprio per come è strutturato. Va perciò bene che ci sia un fondo dal quale devono emergere

l'attenzione per i temi legati al disagio delle persone e dei giovani e gli interventi che sono stati fatti sulla scuola. Ho trovato sinceramente un po' fuori luogo alcuni interventi sull'autonomia differenziata, che forse in questo momento non erano attinenti. come dicevo prima - anche ascoltare interventi che non ci sembrano perfettamente centrati fa parte del confronto che in questa Aula deve avvenire ed è un momento di crescita.

Grazie a tutti. che verranno grazie alle scelte fatte possano aiutare davvero - e sono convinta che aiuteranno - le famiglie, le imprese

stessi relatori hanno sottolineato il problema dei tempi, su cui non tornerò, perché è stato detto in modo chiaro. Voglio, però, dire una cosa. Il senatore Malan ha detto che abbiamo superato tutti i *record*, ma non è così.

mance e altro. Per quello che mi riguarda, vorrei che si scrivesse e si scolpisse nella roccia che non c'è spazio nella legge di bilancio per interventi puntuali, specifici, localistici.

le assunzioni per le Forze dell'ordine, per la Polizia e per i Vigili del fuoco. Quel fondo è servito, in accordo con il Governo, a dare una risposta strategica. E tutte le volte che sento

è perché la scelta più significativa l'abbiamo fatta con le risorse parlamentari, insieme e in accordo con il Governo. Se per la scuola abbiamo risolto il problema del personale ATA e riconosciuto un minimo di risorse per garantire che anche gli insegnanti fossero fossero parificati, nei livelli salariali, al resto della pubblica amministrazione, è perché abbiamo utilizzato le risorse del fondo parlamentare e l'abbiamo fatto insieme. Va bene mettersi gli scudetti sul petto - la politica ha anche questa caratteristica - ma, quando si fa un lavoro comune,

Il fatto che nella manovra di bilancio, per la prima volta, ci siano i livelli essenziali di assistenza è un merito che, *in primis,* dobbiamo riconoscere al Governo perché

di Fratelli d'Italia. C'è un intervento non risolutivo, ma che comunque dà la possibilità di evitare il pagamento dell'IVA che, con un provvedimento recentissimo, in relazione a un'emergenza una questione di rapporti con l'Unione europea - si era introdotto. Sul terzo settore dovremmo riordinare la legge, che

ci sono questioni che non abbiamo trattato e che invece andavano affrontate. Una di queste, collega Floris, è la questione di Air Italy, su

che tutte le compagnie, e non solo Alitalia, ma anche Blue Panorama, Emirates, anche Norwegian e Air Italy hanno avuto la cassa integrazione per il 2022. Qui non potevamo farlo, collega Floris. Anche il Gruppo cui appartengo aveva presentato un emendamento in tal senso, ma non potevamo farlo.

come ha detto il senatore Verducci e ha ragione - i lavoratori dello spettacolo, dell'arte e della cultura sono tra le figure che in questo Paese hanno ricevuto meno anche nell'emergenza Covid e richiedono di più. Su questo dobbiamo cominciare a lavorare, onde evitare che poi ci sia sempre qualcuno in quest'Aula a spiegarci com'è la realtà del Paese. Non siamo disconnessi: sappiamo qual è la realtà del Paese, o meglio, dovremmo saperla.

scrivere con chiarezza in norma primaria che il *payback* si deve pagare interamente, senza sconti, perché per il periodo 2019-2020 vale oltre 2,3 miliardi, che sono fondamentali per reggere l'urto pesantissimo dal Covid. Abbiamo fatto un altro provvedimento per rispondere a quei temi, colleghi, e qui non c'è nessuno che si mette lo scudetto nel petto. Vedete la differenza? Noi abbiamo fatto un provvedimento che consentirà,

evitare così che vadano in piano di rientro e aumentino le tasse. Queste sono misure importanti che, con tutte le nostre difficoltà,

Per fortuna, a fronte della crisi della democrazia che stiamo vivendo, le abbiamo fatte insieme. Riconosciamo in modo comunitario

i tecnici, i tanti vituperati tecnici. E questo voglio dirlo, perché ci sono delle vulgate che dovremmo smentire.

è stato un lavoro veramente grande. Ora valorizziamolo per quello che è, senza parlare di miracoli, perché nessuno ha fatto miracoli, e facciamoci carico di quello che non abbiamo risolto.

più accorato è sicuramente quello della compressione dei tempi. È quello che fa più male a quest'Aula, a tutto il Parlamento e al Governo stesso, che è stato costretto a comprimere così tanto i tempi. Concordo con la relatrice Rivolta. La ricchezza del Parlamento e dei membri delle Commissioni è l'unica risorsa che permette di arrivare fino all'ultimo Comune, all'ultimo territorio di questo Paese, ed è quello che ci permette di fare le scelte, in un modo o nell'altro, ma nel modo corretto. Forse il *record* è stato quello di aver operato, sì, in pochi giorni, non più di quattro, cinque giorni, ma anche con una maggioranza così ampia, una maggioranza che forse questa Repubblica non ha mai visto, e che ha obbligato la stessa maggioranza ad allargarsi ancora di più, anche alle opposizioni, in uno sforzo più grande di se stessa e più grande delle ideologie dei singoli partiti, il che ha aiutato anche il Governo a collaborare in alcune partite importantissime. Senza questa collaborazione alcune risorse non sarebbero mai bastate. Quindi, lo abbiamo fatto insieme, ognuno con la propria parte di risorse a disposizione. Io spero che sia l'ultima manovra

esserci un ritorno alla normalità economica e sociale del Paese, senza dover intervenire d'emergenza e con regole d'emergenza, che oggi hanno la necessità di essere riprogrammate in una normalità anche dal punto di vista normativo. Questa è stata un'altra fatica: faccio una norma d'emergenza o faccio una norma strutturale? Quante volte ce lo siamo chiesti nelle ultime settimane? Il rallentamento è dovuto anche al fatto che raggiungere l'obiettivo dei 51 obiettivi del PNRR era difficile. Ma è stato raggiunto ed è stato raggiunto con la decretazione d'urgenza, che ha ancor di più compresso tutti quelli che sono i tempi del Parlamento. Abbiamo lavorato ancora una volta con un metodo che da qualche anno vediamo, quello dei temi comuni, che ha permesso alla maggioranza di mettere insieme risorse che separatamente non avrebbe avuto. Una volta non si faceva così: si prendevano le risorse del Parlamento e i parlamentari le dividevano. A chi

per l'autismo e il bullismo. Insomma, penso a tutti quei fondi che qualcuno potrebbe ritenere secondari e che, invece, danno delle risposte a un Parlamento, sì compresso, ma che sa benissimo che anche un fondo da 5 milioni fa la differenza.

anche numericamente. Gli Uffici ci hanno sostenuto e lo hanno fatto veramente con tutta la voglia di sorreggere lo sforzo della macchina dello Stato. Così è stato tutti i giorni. Non era semplice. Forse, se non fosse arrivato il Natale, ci avremmo messo qualche giorno in più, ma non si poteva fare diversamente. Mi auguro davvero che questa sia l'ultima manovra